L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 30 luglio. Nella seduta odierna proseguirà la discussione generale sul disegno di legge sul contrasto della discriminazione o violenza per sesso, genere o disabilità. L'ordine del giorno della seduta di domani, con inizio alle ore 9,30, prevede la discussione del decreto-legge in materia di imprese, lavoro, giovani e salute. Orientativamente intorno alle ore 11,30 il Ministro della giustizia renderà un'informativa sui gravi fatti occorsi nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. I Gruppi potranno intervenire per dieci minuti, divisibili in due interventi minuti al Gruppo Misto, divisibili in tre interventi). Al termine dell'informativa la seduta sarà sospesa per la sanificazione dell'Aula. Alla ripresa, alle ore 16,30, proseguirà la discussione del decreto-legge in materia di imprese, lavoro, giovani e salute. Poiché il Governo ha preannunciato la posizione la posizione della questione di fiducia sul decreto, nella serata di domani sarà convocata una Conferenza dei Capigruppo che definirà le successive fasi procedurali di esame del provvedimento, da svolgersi nella giornata di giovedì 22. Sempre nella giornata di giovedì 22, alle ore 15, si svolgerà il *question time*, con la presenza dei Ministri dell'interno, della difesa e del lavoro. Il calendario della prossima settimana prevede, con sedute a partire dal pomeriggio di martedì 27 fino a venerdì 30 luglio, se necessario, la discussione dei decreti-legge *governance* PNRR e semplificazioni, attualmente in corso di esame presso la Camera dei reputati, e rafforzamento pubbliche amministrazioni e giustizia. Giovedì 29 luglio, alle ore 15, avrà luogo, come di consueto, il *question time.*

mi domando dunque se si debba intervenire nuovamente sull'atteggiamento da tenere nei confronti dei senatori che decidono di non procedere alla vaccinazione e se ci siano interventi possibili.

personalmente sono vaccinato e credo che lo sia gran parte dei senatori, ma, visto che pone il problema, le do subito la mia opinione personale:

delle cosiddette minoranze e chi invece le vuole opprimere o mettere il tallone sopra i loro diritti. Non è assolutamente così! Capisco che il segretario del Partito Democratico si trovi nella condizione in cui si è trovato qualche altro segretario

le critiche che venivano da più parti, non soltanto dal centrodestra e dalla destra, ma da tutto lo schieramento politico e da personalità che vengono dal mondo *gay* e lesbico e dal femminismo. Niente: non ha voluto ascoltare alcunché e ci porta

Il pensiero che c'è dietro l'azione politica di Letta, è ben altro: non è la difesa degli omosessuali o delle persone che si sentono discriminate. Non è questo il problema di Letta, è ben altro: far passare altri messaggi e svolgere una battaglia politica in cui, a questo punto, gli omosessuali sono una sorta di specchietto per le allodole, qualcosa da utilizzare per fare una campagna politica ben definita per raggiungere determinati ambienti, anche estremisti, su questi temi a cui si strizza l'occhio. Al contrario, non si ha in mente l'obiettivo finale, che dovrebbe essere quello di salvaguardare le minoranze e tutelare chi è discriminato.

del centrosinistra. Lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle in anni lontani, come ricordava Ignazio La Russa qualche giorno fa proprio su questo tema in quest'Aula. Mi riferisco alla discriminazione da parte di vostri fratelli, probabilmente vostri padri politici in quegli anni, che discriminavano chi non la pensava come loro: ci siamo visti allontanare dalle scuole e dalle università; ci è stata sottratta la possibilità di entrare in quei posti soltanto perché avevamo il marchio, perché avevamo il marchio, eravamo di destra e venivamo classificati e chiamati in un determinato modo; non avevamo udienza in quei posti. Abbiamo sentito sulla nostra pelle che cosa significava essere discriminati ed essere nella condizione di non partecipare e di non essere uguali agli altri, anche se poi gli spazi ce li siamo presi lo stesso, sia chiaro.

giornale o la televisione e che vediamo pontificare sul fatto che non si debba discriminare nessuno e si debba essere tolleranti. In quegli anni non erano tolleranti, non lo erano con noi. Dirò di più: provengo da

e di avere amici che avevano tendenze sessuali diverse: anche loro venivano discriminati in quel mondo, perché in quegli anni succedeva questo, e non stiamo parlando di ottant'anni fa, ma di quaranta. Erano anni in cui la sinistra diceva determinate cose, si comportava in un certo modo e aveva

non solo. Abbiamo anche visto - sempre in ordine a questo tema - che ultimamente il segretario Letta chiede al nostro *leader* di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni di prendere le distanze da

che dietro questo disegno di legge c'è ben altro: un percorso di carattere culturale che viene proposto alle giovani generazioni; la teoria *gender* da propagandare all'interno delle scuole; il principio che debba essere respinta la sessualità biologica, per cui non devono più esserci un uomo e una donna, ma semmai si deve passare all'identità sessuale percepita, con tutte le problematiche che questo comporterebbe in tanti ambienti. Ci sono

nelle piazze, anche attraverso un *referendum*, per fare in modo che questa legge liberticida non passi e non sia una legge dello Stato italiano. *(Applausi.

l'intendimento e il luogo comune che si vogliono creare. Se un cittadino italiano o un parlamentare della Repubblica dice di essere per la famiglia tradizionale, immediatamente viene bollato come omofobo e si sentono voci che vogliono dipingere questa opinione come fascismo.

coloro che si permettono di assumere atteggiamenti che il nostro codice già colpisce. Nessuno in Italia, che è un Paese civile, può permettersi di aggredire o discriminare senza motivo qualcuno. Fratelli d'Italia ha detto chiaramente c'è piena disponibilità, come sempre, ad affrontare con inasprimento di pene ogni fenomenologia che si dovesse accentuare nella nostra società, società, perché viviamo in uno Stato di diritto. Cosa diversa, invece, è quello che la sinistra

identità e di consenso che evidentemente vive nella nostra Nazione proprio per un distaccamento totale dal mondo reale. Saremo in quest'Aula per settimane a parlare di ciò,

nella difficoltà di una crisi economica che era già evidente prima della pandemia e che l'emergenza sanitaria ha reso estrema, con infinita incertezza per il futuro. Dobbiamo parlare invece della legge Zan: è questa la priorità delle priorità, che dimostra plasticamente, anche su questo,

Noi non accettiamo nessuna possibilità di compromesso. Nonostante ciò, come siamo stati abituati dal nostro *leader* Giorgia Meloni, cerchiamo di fare un lavoro serio per il rispetto che abbiamo degli italiani e dell'alta istituzione che rappresentiamo. Fratelli d'Italia ha presentato 127 emendamenti e sei ordini del giorno, che sono le nostre proposte per smantellare questo provvedimento ideologico sbagliato e per noi pernicioso per la società, senza mediazione, perché, al cospetto della furia ideologica che viene messa in campo, non si può avere altro atteggiamento. Peraltro - come viene confermato dall'atteggiamento della sinistra nei confronti dei suoi alleati della maggioranza - anche quello che è avvenuto dal punto di vista istituzionale è estremamente grave. Senato è stata trasformata nella Commissione, la quale invece è stata completamente esautorata della sua funzione. agli italiani: «Siete liberi di pensare, a condizione che non diciate». È il tipico atteggiamento della sinistra, che pensa di avere la verità in tasca e di essersi trasformata nella motorizzazione civile che rilascia le patenti di civiltà a chi la vuole pensare diversamente. Il collega Totaro lo ha detto in maniera molto chiara chiara e netta. Non ci impressioniamo e siamo fortemente supportati da quello che raccogliamo, stando ogni giorno nelle piazze. Abbiamo animato centinaia di gazebo già negli scorsi fine settimana e questa legge non ha l'approvazione non soltanto di quest'Aula, ma soprattutto dei cittadini italiani, che hanno capito che si vuole fare altro, ossia mettere un bavaglio e capovolgere una discriminazione,

legittima ed espressa magari in forme consone. Non ci fermeremo con quest'attività di confronto con i cittadini; metteremo in campo ogni azione politica per dire, come come ha fatto il presidente La Russa nel suo intervento, che non si può promuovere l'odio nel nome dell'amore.

siamo in quest'Aula a confrontarci ancora in una discussione su un argomento particolarmente divisivo. Personalmente, lo trovo un dibattito veramente democratico su un argomento che però, in una scala di priorità, per me non è al primo posto, come potrebbero essere invece tante altre questioni da risolvere nel nostro Paese. Tanti altri provvedimenti sono passati velocemente, quasi in sordina, eppure, quelli sì, avrebbero avuto bisogno di essere dibattuti a lungo in quest'Aula prima dell'approvazione definitiva. provvedimenti che vanno a limitare le libertà fondamentali garantite dalla nostra Costituzione. Ad esempio, abbiamo dibattuto sommariamente sulle strategie per combattere il covid: tutti sappiamo che la vittoria su di esso è fondamentale per tornare ai diritti di libertà che ci sono stati negati. Il dibattito sulle cure domiciliari precoci si è limitato a un voto su una mozione, che poi è rimasta per ora lettera morta. Perché quella vaccinale dev'essere l'unica strategia? Perché non si affianca quella delle cure

questa sì che è una discriminazione vera e propria. Torniamo però al disegno di legge Zan e al suo boicottaggio in Commissione, come affermano i sostenitori - dico io - in malafede. Tanti sono i provvedimenti fermi. Cosa dobbiamo dire, ad esempio, del disegno di legge n. 189 sui disturbi del comportamento alimentare? Parliamo del serio problema dell'anoressia e della bulimia grave, soprattutto tra i giovani. È fermo dal marzo 2018.

n. 992, sull'insegnamento dell'educazione motoria nelle scuole primarie, riguarda un argomento cui tengo particolarmente, perché fare sport correttamente fin da bambini fa crescere adulti in salute ed equilibrati, ma questo per molti di voi colleghi

sulla prevenzione dei maltrattamenti a danno di minori e anziani disabili attraverso l'istallazione nelle strutture di telecamere di videosorveglianza, già approvato alla Camera il 23 ottobre 2018 e bloccato miseramente in Senato. Noi di cosa stiamo parlando? *(Applausi)*. Stiamo parlando di un provvedimento che pone l'attenzione su una categoria sicuramente fragile e che va tutelata, ma come tante altre. Qual è il discrimine che vi porta a dire che è più importante tutelare e proteggere dalla violenza un transessuale, un anziano in una casa di cura o un bambino in un asilo? Signor Presidente, perché l'emiciclo alla sua sinistra si scandalizza tanto, fa tanto rumore e forza la mano con gli alleati di Governo su un provvedimento fermo in Senato da qualche mese e non si scandalizza per un provvedimento contro la violenza su bambini e anziani fermo in Senato da anni? *(Applausi)*. Forse anziani e bambini hanno per loro meno importanza rispetto al mondo votante di lesbiche, *gay*, bisessuali, transessuali e transgender (LGBT)? La violenza è sempre tale e sempre da condannare, che si tratti di una persona adulta, anziana o minore di qualsiasi tendenza sessuale. ovvio che esistono delle fragilità che vanno maggiormente tutelate, ma non con questa legge che, dietro la facciata illusoria della tutela, presenta molti aspetti problematici. È scritta male. Abbiamo già tante restrizioni che ci condizionano e non possiamo aggiungere una legge che mette il bavaglio su alcuni argomenti di opinioni e sensibilità personali. I bambini hanno bisogno di crescere sereni con una mamma e un papà, che naturalmente sono donna e uomo, con le loro tipiche caratteristiche biologiche, fisiche e attitudinali, che sono diverse per natura. Questa è un'affermazione che potrebbe urtare la sensibilità di un appartenente alla categoria LGBT e magari mandare a giudizio qualcuno. Un aspetto di questo disegno di legge che mi urta particolarmente è legato alle conseguenze che può avere nello sport femminile. Da ex ciclista agonista devo ritenermi particolarmente fortunata per aver svolto la mia attività negli anni Novanta. Infatti, nei Paesi in cui queste norme sono già attive si stanno oggi verificando casi di prevaricazione da parte di uomini che, sentendosi donne, scippano le medaglie alle donne. qualche esempio. Cristina Sanulli e Denise Neumann sono due atlete che hanno saputo costruirsi, ovviamente a prezzo di duri sacrifici, un percorso di eccellenza sportiva nel panorama dell'atletica leggera, riuscendo a conciliare il lavoro, lo sport e gli impegni familiari. Erano imbattibili e, tuttavia, a fine 2020 sono state costrette a lasciare la medaglia d'oro a Valentina Petrillo, atleta transgender uomo che si percepisce donna. Un altro esempio è Rodrigo, che è un lui, una lei nato nel 1984, alto 1,94 metri e che fino al 2015 ha giocato nei campionati maschili di pallavolo. Da quell'anno si fa però chiamare Tiffany. Per carità, nulla da osservare, ma il punto è che nel 2017 ha esordito nel campionato femminile italiano, giocando con il Palmi per una stagione. Ora gioca nella nazionale brasiliana femminile di pallavolo e probabilmente parteciperà alle prossime Olimpiadi di Tokyo. La sua statura e i suoi muscoli maschili hanno preso il posto di un'atleta femmina che magari ha passato anni ad allenarsi per poter giocare alle Olimpiadi nella squadra femminile. è rappresentato da Laurel Hubbard, un signore di mezza età, nato Gavin, che da ragazzino aveva la passione per il sollevamento pesi. Si era classificato primo in un concorso *junior* del 1998, ma poi non aveva più vinto nulla. c'è stata la svolta: dopo aver deciso di diventare donna, ha cominciato a gareggiare nelle competizioni femminili. Poiché ha vinto tutto (quindi togliendo alle atlete donne la vittoria), rappresenterà la Nuova Zelanda nelle gare femminili delle prossime Olimpiadi di Tokyo. anche a Gabrielle Ludwig, un signore sulla cinquantina, muscoloso e alto due metri, che si sente donna. E fin qui nessun problema, per carità: ognuno nella vita è libero di fare un po' come crede. Tuttavia, dal 2013, in base alle norme americane scritte sotto dettatura delle *lobby* LGBT, Ludwig gioca a *basket* nel campionato femminile studentesco. Le sue compagne di squadra ovviamente lo adorano, ma le avversarie un po' meno. Colleghi, vi rendete conto delle aberrazioni a cui si andrà incontro approvando così questo disegno di legge? Un altro aspetto che mi inquieta è legato a scuole e bambini.

o, al limite, i ragazzi a partire dalla pubertà? I bambini hanno bisogno di imparare il rispetto - quello sì - ma verso il prossimo e tutte le diversità.

che sento è il continuo attacco politico alle nostre idee, la supponenza tutta di sinistra di essere detentori detentori della verità, gli ingiustificati atteggiamenti di superiorità da parte di alcuni. Mi sento discriminata quando un collega o una collega non risponde al mio saluto soltanto perché ho un'idea diversa dalla sua. lui o lei pensa che sia così. Colleghi, il rispetto parte da qui: dal rispetto tra di noi, dal rispetto per le idee di tutti; non è mettendo un bavaglio

su cui procedere. Credo di poter dire che in Aula abbiamo trovato parecchio consenso, anche perché i principi sui quali noi viaggiamo sono sempre quelli della libertà Quando si devono affrontare argomenti così delicati, è sempre necessario far precedere gli incontri, i dibattiti, gli interventi in Aula da confronti, devo ringraziare la presidente del nostro Gruppo, Anna Maria Bernini *(Applausi)*, per aver consentito al nostro Gruppo di affrontare questo argomento estremamente delicato con quella necessaria saggezza che occorre e con quel buon senso che credo caratterizzi un movimento politico come il nostro: quindi nella sua assoluta libertà, ma nel rigore e nel rispetto di quei valori, soprattutto di libertà e di democrazia, che sono tipici dei movimenti politici che hanno qualcosa da dire anche in termini di civiltà. di civiltà. Prima di fare questo intervento, mi sono domandato tante volte a quali valori avrei fatto riferimento. È la vita di ciascuno di noi che ci porta in momenti delicati come questi a fare un po' il riassunto della propria vita. Allora tornano alla mente i principi e i valori, quelli che ci sono stati consegnati non solamente ai tempi della scuola, ma anche a chi ha frequentato la parrocchia, a chi ha avuto la ventura di vivere soprattutto in una famiglia che ha donato qualcosa, come hanno fatto i miei genitori che hanno sempre messo al centro e mi hanno insegnato il rispetto della persona, soprattutto il rispetto della dignità

lungo il marciapiede - ciascuno di noi continua a essere militante di un partito politico - ci si trova inevitabilmente a doversi confrontare con coloro che incontriamo, che firmano

dopo la domanda di rito «Che cosa si dice a Roma» - è una di quelle domande aperte alle quali è difficile dare una risposta, ma immagino che a ciascuno di voi sul territorio accada ed è forse una delle più insidiose - la prima cosa

di questa maggioranza. È una maggioranza nata nella necessità di fare qualcosa per l'Italia. Questo è un Governo più che di solidarietà nazionale, di necessità nazionale, e deve affrontare due temi primari.

- bisogna mettere al centro le cure. Noi dovremmo mettere al centro della nostra battaglia e del nostro impegno politico innanzitutto la cura contro questo mostro maledetto e, per farlo, dobbiamo porre il problema della sanità tra quelli principali. La stessa cosa vale per l'economia: in un momento in cui abbiamo la necessità di tirare fuori l'Italia dalle sabbie mobili; nel momento in cui rischia di arrivare la disoccupazione, quella vera; in un momento in cui le tensioni sociali potrebbero arrivare al culmine, noi noi abbiamo un Presidente del Consiglio che giustamente ha detto che questo è il momento di dare e non di togliere; questo è il momento di rilanciare l'economia. Allora, economia e tentativo di sconfitta del Covid-19 sono Invece siamo arrivati qua. Non voglio iscrivermi al partito del benaltrismo - figuriamoci, in tanti ci sono già - ma mi pare che in questo momento un tema così divisivo dovrebbe essere trattato in maniera estremamente delicata. Colleghi, non la pensate magari come la penso io o come la pensano tanti colleghi, ma avremmo la possibilità - basta poco, forse poche ore, pochi giorni immediatamente e sotterrare quell'ascia di guerra che qualcuno ha tirato fuori, evitare di parlare - come si diceva una volta nei film western - con lingua biforcuta e andare al al sodo, guardare quali sono i problemi. Allora, se si deve risolvere un problema, perché c'è un *vulnus* nel nostro ordinamento, proviamo a metterci d'accordo, proviamo a trovare una soluzione. Qui pare invece che si voglia arrivare ad affossare tutto, perché si arriverà al voto segreto e incominceranno a cadere alcuni emendamenti. Quello che qualcuno voleva portare a casa, l'asticella messa al minimo, non arriverà. Allora, siccome molti di voi stanno pattinando su una lastra di ghiaccio estremamente sottile, invito alla ragionevolezza e alla calma.

non siamo di fronte alle Tavole della Legge. Siamo di fronte a un provvedimento che sicuramente può essere migliorato se semplicemente uscisse dalle categorie di certo fanatismo che abbiamo visto anche in quest'Aula. Quello che vi voglio dire è che anche il Partito Democratico ha commesso un grave errore. Il rischio è quello di vederlo indirizzato verso una direzione chiara: diventare la sesta stella dei grillini. Questo è un problema dal quale dovreste provare a venire fuori. Certamente, capisco tutto, i ragionamenti legati alle alleanze, ma è possibile che il segretario Enrico Letta del Partito Democratico come primo provvedimento, tornato dalla Francia, abbia parlato di *ius soli*, di disegno di legge Zan, di patrimoniale e poi ancora - com'è avvenuto qualche giorno fa - di tassa sulla successione?

Questo è avvenuto. Capisco anche il tentativo che avete fatto per provare a rendere più edulcorata la pillola, narrando che è stato opportuno inserire il termine "disabilità". Ma, se noi andiamo a guardare il provvedimento, ci rendiamo conto non solamente che questa legge è stata scritta male, che la disabilità compare in un solo articolo - non c'è, ad esempio, nell'articolo 1 - e che comunque dovremmo chiarire cosa si intende per disabilità. È l'invalidità

(in particolare nel penale), che il nostro ordinamento contempla tutto quanto è necessario per evitare che comportamenti discriminatori si possano verificare e non lo dico soltanto io, ma lo dicono tutti - nel rispetto del principio previsto dall'articolo 3 della nostra Carta costituzionale, al quale questo provvedimento è

controfirmato dal Presidente della Repubblica, posto che è contrario non solamente all'articolo 3, ma anche all'articolo 21 e a buona parte degli articoli della Costituzione.

che lei si è rivolto al mio partito, dicendoci di fare il Partito Democratico e non la sesta stella. Vede, senatore Aimi, forse a lei sfugge che là dove ci sono i diritti, dove c'è il rispetto degli altri e dove c'è l'accoglienza, il Partito Democratico c'è sempre stato, c'è ancora e ci sarà sempre. E questo è nei valori e nelle radici del Partito Democratico. Non ci insegni dove stare, senatore Aimi: sappiamo perfettamente cosa siamo e cosa vogliamo. Per esempio, in merito a questo disegno di legge, legge, vedo che c'è una narrazione e c'è una realtà. La narrazione è composta di tanti elementi e ad essi proverò a ribattere, uno per uno, essendomi concentrata soltanto su alcuni.

Io non so, cari colleghi e care colleghe, se voi avete una concezione di voi stessi così bassa da non essere capaci di tenere insieme i provvedimenti di cui il Paese sicuramente ha bisogno in questo momento momento e altri tipi di provvedimenti, come il disegno di legge in esame, che vuole tutelare persone che ogni giorno si svegliano e pensano di non andare bene all'Italia nel 2021. nel 2021. Vi chiedo: siamo capaci di rispondere a queste necessità? Io penso proprio di sì. Voi dovete rispondere a questo, perché richiamare sempre il fatto che siamo occupati in altro non rende giustizia a una grande parte del Paese che ogni giorno si sveglia e sente di essere sbagliata. E questo non ce lo possiamo permettere. Sento dire in quest'Aula che il provvedimento sarebbe divisivo. Mi chiedo per chi sia divisivo e mi rispondo: per chi vede la diversità come un problema.

che amino persone dello stesso sesso, che non si trovino nel corpo in cui sono nate. Allora, cari colleghi e care colleghe, vi chiedo: per chi è divisivo? Mi do la è divisivo per chi non accetta l'altro, per chi non ha rispetto dell'altro. Il Partito Democratico su questo sa da che parte stare. *(Applausi)*. Ho sentito tante volte dire in quest'Aula che l'articolo 4 del provvedimento limiterebbe la libertà di espressione. Su questo si si potrebbe rispondere molto velocemente. Infatti, se chi lo afferma ne è convinto, o mente sapendo di mentire oppure afferma che in questo Paese da trent'anni la libertà di espressione su certi temi

che le persone possano esprimere esattamente e liberamente quello che sono? La libertà di espressione è stata assolutamente tutelata - pensate - persino quando qualcuno ha detto «chiudiamo i porti».

del grido «al lupo, al lupo, attenzione all'orco! Qualcuno pensi ai bambini». È vero, è la famiglia, il primo nucleo fondamentale della società, che deve garantire l'educazione dei figli;

dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni». Colleghi e colleghe, anche i genitori hanno l'obbligo morale di assistere i loro figli, che non possono sentirsi sbagliati, non possono aver paura di sentirsi

Si richiama più e più volte la narrazione secondo la quale c'è un orco che vuole portare via i nostri figli, che li vuole educare in un certo modo, ma questo è quanto di più falso. E allora, cari genitori che siete in quest'Aula, provate anche voi a a fare attenzione alle inclinazioni dei vostri figli, che non devono avere paura del mondo in cui vivono. In Italia, nel 2021, si deve far sì che ciascun figlio e ciascuna figlia possano essere liberi di essere quello che Ho sentito dire in quest'Aula che la mattina ci si può svegliare alberi e ci si può addormentare uomini, che ci si può svegliare donna se si è uomo e ci si può addormentare in un altro modo. Non è così. Anche in questo caso diciamolo chiaramente. Abbiate il coraggio di dire che non vi sta bene questo disegno di legge e non lo volete approvare.

Possiamo avere varie interpretazioni e idee sull'identità di genere - cari colleghi e care colleghe - anche sulle estremizzazioni che questo concetto porta con sé, ma ci sono migliaia di persone che ogni giorno si svegliano e non stanno bene nel corpo che hanno. Noi, come legislatori, siamo tenuti a considerarlo, a dare loro una risposta, perché per questo vengono picchiati, vengono odiati, vengono discriminati. Sono stati fatti anche tantissimi esempi, ciascuno di noi ne può fare. Ne ho sentiti dei più strani, dei più mostruosi intorno a questo argomento, ma ciascuno di noi ne può fare. Non fanno statistica gli esempi. Io vi potrei fare nomi di decine e decine di persone, amici e amiche carissime, che vivono e hanno vissuto giornalmente la paura, la discriminazione, il fatto di non poter vivere liberamente. Se questo a voi sembra normale, mi chiedo che idea avete dell'Italia del 2021.

che ho una storia molto molto precisa e molto particolare che mi ha insegnato esattamente che le persone devono essere accolte, devono essere Io credo, però, che ciascuno di noi qui debba mollare quello che è. Io sono anche molto fortunata, perché sono donna, sono bianca, sono cattolica, sono normodotata e potrei continuare ancora.

però che noi dobbiamo lasciare quello che siamo e provare per tre minuti a camminare nelle scarpe degli altri. Non so se l'avete mai fatto: è un esercizio importante, un esercizio bello. bello. Mi dovete spiegare perché no, perché tutto quello a cui vi siete attaccati in questo dibattito, in questa discussione in cui si è sentito di tutto fuorché, molte volte, la verità, ci dovete dire perché no, perché non volete, nel 2021, in Italia che migliaia di persone si possano alzare e non avere più paura, perché lo Stato non deve poter garantire loro di non avere paura. Il mondo va avanti, colleghi e colleghe, che ci piaccia o meno. Noi possiamo prenderne atto ed essere all'altezza del mondo fuori, oppure continuare a strumentalizzare la vita delle persone.

oltre un anno e mezzo di pandemia nel quale l'emergenza ha stravolto i programmi di Governo, ha dettato nuovi obiettivi, perseguiti con evidenza e in maniera diversa dai due Governi e determinato i conseguenti provvedimenti, ora siamo a discutere un disegno di legge che nulla ha a che fare con i ristori o i sostegni, con la cassa integrazione, le proroghe, gli incentivi per una auspicata ripresa, le risorse per i vaccini, le cure sanitarie. Coniugare l'emergenza e l'ordinarietà si può fare, dipende come, ovviamente. Ora ci troviamo a parlare di diritti civili.

"Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità". Il titolo ben ci predispone, salvo poi, all'articolo 1, definire in modo arbitrario tali categorie e lasciare ampi margini di discrezionalità. Una attenta analisi del testo ha fatto emergere insidiose criticità, che sono state rilevate

il già citato Giovanni Maria Flick e da tanti altri auditi, e, non ultima, dalla preoccupazione espressa dal Vaticano. Una legge deve essere fatta bene, tenendo conto delle conseguenze che può avere a 360 gradi, non adducendo ad ambiguità che delegherebbero ai giudici non l'applicazione della legge, ma la sua interpretazione. Quando, all'articolo 4, si parla di libertà di espressione, «purché non idonea a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti», chi deciderà l'entità di questo concreto pericolo? Chi determinerà l'ambito in cui l'opinione diventa minaccia e odio o quello in cui l'opinione resta espressione di un punto di vista? Sono confini non definiti, parametri inesistenti che rischiano tanti bavagli e tanti processi. Questo provvedimento, così come è stato scritto, persegue le idee e l'espressione delle stesse prima dei comportamenti, e questo per noi è inaccettabile. È vero: questo disegno di legge è stato approvato alla Camera dei deputati. E allora? Esistono proprio per questi motivi le due Camere. Esiste ancora il bicameralismo perfetto, nonostante in questa legislatura, anche prima della pandemia, sia stato continuamente affossato a colpi di fiducia, anche quando l'emergenza non era una prerogativa. Esiste ancora e lo hanno deciso gli italiani votando al *referendum* nel 2016. Esiste ancora, nonostante continue sferzate per affossarlo: l'ultima, il voto per il Senato ai diciottenni. Allora, se il bicameralismo esiste, non permettere al Senato di apportare modifiche a un provvedimento in discussione sarebbe addirittura incostituzionale. Poter correggere un testo, poterlo modificare per migliorarlo e ottenere così una maggiore condivisione, soprattutto in questo Governo di unità nazionale, dove una maggioranza composita sta trovando delle convergenze con l'unico obiettivo di portar fuori il Paese dalla crisi, significa non demolire un disegno di legge, ma imprimergli una forza maggiore, dando il giusto rilievo ai temi trattati. È evidente che il disegno di legge Zan, così concepito, divide il Paese a metà. Divide questo Parlamento a metà. Perché, allora, non provare a migliorarlo? Dispiace constatare che a certa parte politica interessi più poter mettere la propria bandierina e ideologizzare il provvedimento, piuttosto che affrontare il confronto per dare, tutti insieme, un voto favorevole alla lotta contro l'omotransfobia; una battaglia che deve non dividere, ma unire; che deve non degenerare i forti contrasti politici dentro e fuori il Parlamento, ma perseguire una dialettica anche accesa, ma sempre all'insegna del rispetto. *(Applausi)*. che sempre più spesso sparisce dal vocabolario, ma che in realtà dovrebbe tornare ad essere la parola chiave, sempre e in qualsiasi situazione, è veramente dimenticata. Quando si parla di rispetto nelle scuole, questo non deve poter essere confuso con la teoria del genere e di ogni forma educativa all'orientamento sessuale; prerogativa, questa, della sovranità educativa della famiglia. Non "anche i genitori hanno il diritto di seguire moralmente le inclinazioni naturali dei propri figli": loro hanno il diritto di farlo. La scuola, infatti, non può sostituirsi alla famiglia, perché si travalicherebbe la libertà dell'individuo, ovvero la libertà dei nostri bambini. POF e programmi condivisi con i genitori non possono essere uno strumento che ne assicura l'esclusione. L'insegnamento di certe teorie nella scuola non deve essere consentito a priori, in maniera chiara. Aprire e non chiudere: questo è quello che chiediamo. Le barricate ideologiche non portano a nulla di buono. Vogliamo difendere i diritti di tutti e combattere ogni forma di violenza, ma lo vogliamo fare in maniera efficace, scrivendo una legge in modo chiaro, che esprima la volontà del legislatore e non quella di chi la deve interpretare. In base ai nostri valori e alla nostra cultura liberale, condanniamo ovviamente qualsiasi discriminazione e qualsiasi manifestazione d'odio nei confronti di qualunque essere umano, titolare per definizione della propria altissima e intoccabile dignità. Per questo motivo e per adempiere al mandato del Governo, che convintamente sosteniamo, siamo stati e siamo quindi disponibili a concordare delle modifiche che ci permettano di votare questo provvedimento. C'è una questione di fondo, però, che mi preme evidenziare. Proprio per la nostra cultura e i nostri valori, crediamo fermamente che tutti i cittadini abbiano gli stessi diritti e non che vi siano alcuni che abbiano diritti che prevalgano rispetto ai diritti di altri. altri. Questo provvedimento, come molti provvedimenti di matrice culturale di sinistra, è basato sulla categorizzazione dei cittadini, creando proprio per questo discriminazione tra categorie ed esclusione di alcuni rispetto ad altri. Con l'approccio per categorie, le casistiche che si vengono pertanto a creare per ricomprendere tutti sono innumerevoli, quasi infinite, perché innumerevoli e infinite sono le caratteristiche dei cittadini, in quanto esseri umani. Non è certo inserendo la categoria dei disabili che, tra parentesi, con l'orientamento e il genere sessuale non c'entra proprio niente, che si è risolto il problema. *(Applausi)*. È proprio l'approccio che è sbagliato. Basando invece i provvedimenti legislativi sulla considerazione del rispetto per tutti i cittadini, come titolari di pari dignità e di pari diritti, di pari livello, non si crea discriminazione e anzi vi si pone rimedio. signor Presidente, se l'obiettivo dichiarato di contrastare le discriminazioni e l'istigazione all'odio era condivisibile e lodevole, legge Zan, intransigente e rigido, con cui si vuole perseguirlo, risulta evidentemente provocatorio, se non controproducente.

in Aula del disegno di legge in esame partendo da un presupposto diverso, anche se è stato più volte menzionato da parte di altri colleghi: l'etica. Non penso si possano affrontare argomenti così delicati, come quello della sessualità in tutte le sue forme e sfumature,

diverse peculiarità che ciascuno di noi porta in sé e che fanno di ciascuno di noi il proprio essere. Sono diversa dalla collega Rivolta o dal collega Centinaio: siamo tutti diversi, ma non solo per il per il nostro genere sessuale. Siamo diversi perché siamo composti così diversamente per come pensiamo, per come sentiamo. È come se volessimo cercare di disciplinare il concetto di fede

Quello di fede è un concetto altamente personale, appartiene alla persona; non per questo non è discriminato. Chi è cristiano è stato perseguitato e lo è tuttora; chi è musulmano ha un'idea totalmente diversa, chi è buddista non riconosce. Abbiamo mille forme. Lo stesso discorso vale per il dolore: come si fa a disciplinare la soglia del dolore? Un medico - ho una figlia medico - ti

che sicuramente sarà discriminato; è normale, anche qui ci sono le discriminazioni, fanno parte della vita. Personalmente non me la prendo, è tutta esperienza: più si viene discriminati, più si cresce. Purtroppo, sono cresciuta così; non ho alcun problema ad ammetterlo.

così sviscerato nell'ambito del perché e del per come, non entra nell'animo umano che, comunque sia, deve essere sempre preservato, tutelato e soprattutto rispettato. testo dà la possibilità di impostare un progetto di etica nelle scuole, finalizzato a cercare di far capire l'importanza del rispetto del proprio corpo, dell'approccio con gli altri, del rispetto della non violenza, e magari di aiutare i genitori che hanno più difficoltà in questo percorso.

Questo forse cozza con il mio modo di sentire; ripeto, non si possono disciplinare delle sensazioni. Non sono un medico né uno scienziato; non so cosa significhi sentirsi donna in un corpo di uomo e viceversa. Sono nata donna e morirò donna, va bene così *(Applausi)*; mi dispiace per coloro che invece sentono questa cosa per la quale nutro grande rispetto. A me non interessa l'orientamento sessuale:

con coloro che non hanno la fede; può essere puntato il dito nei confronti di chi non è come te. Quindi, in generale, se dovessimo disciplinare tutto lo scibile delle discriminazioni dovremmo mettere da parte le decine di leggi che la senatrice Ferrero ha detto essere ferme e concentrarci solo su questo. E invece dovremmo lasciare andare la nostra natura. La natura ha fatto ciascuno di noi come vuole; siamo sotto la volta del cielo, abbiamo un inizio e una fine, però, certo, dovremmo concentrarci e rafforzare là dove il sistema è debole, cercando di rafforzare l'etica e la certezza della pena,

abbiamo giustizia. Ma non solo con il tormentone sul giornale piuttosto che nelle trasmissioni televisive dove vengono proposti e riproposti nuovamente situazioni e accadimenti che tante volte non sono altro che il pungolo per andare magari a rifare la stessa cosa.

le gabbie - chiamiamole così - come, purtroppo, succede, si è praticamente lasciato andare tutto e improvvisamente abbiamo avuto episodi di violenza all'estremo. Questo forse è un altro degli elementi su cui dobbiamo soffermarci e su cui puntare la nostra attenzione. Non penso che ci sia una legge che il Partito

buonsenso, che questo tema che abbiamo toccato vada oltre il buonsenso, che avere buonsenso significhi legiferare per il rispetto di tutti

da soli potessimo cambiare il nostro sesso e il nostro modo di fare. *(Applausi)*. Invece non siamo così, noi siamo come Dio ci ha fatti e dobbiamo accettarci, non possiamo spingerci oltre, mai spingersi oltre la natura. Va bene aiutarci, disciplinare, ma non andare oltre quello che ci è stato consentito,

La cosa importante è cercare di continuare a considerarci esseri umani, con tutte le nostre sfumature. Ho fatto il sindaco

e lo dico qui con grande orgoglio, a quasi sessant'anni: ho cresciuto una figlia da sola, perché l'uomo - mio marito - che l'ha concepita con me mi ha lasciata che mia figlia aveva sette anni e ce l'ho fatta da sola, con il mio sesso di donna, di madre, senza nessun problema e ne sono orgogliosa.

per loro natura, i fratelli più piccoli guardano alle mode, alle frequentazioni e ai costumi di quelli maggiori e così è stato anche nella mia famiglia, nella mia generazione. Ho un fratello che ha vissuto la gioventù negli anni Ottanta,

Si amavano, all'epoca, David Bowie, Lou Reed, Elton John, Freddie Mercury, George Michael e nessuno si poneva la questione di quali fossero i loro orientamenti sessuali. una generazione che ascoltava e partecipava in massa ai concerti dei Led Zeppelin, senza porsi alcun problema sui testi che oggi sarebbero stati bollati come sessisti. Quando fu la volta di Boy George e di Annie Lennox, nessuno si chiese se a loro piacesse il maschio, la femmina o entrambi. Ci innamorammo della loro musica e delle loro voci: *stop*. Non c'erano solerti commissioni censorie o progressisti di professione a giudicare o a fare proseliti. Ci si appassionava alla loro musica, ai personaggi, senza porsi chissà quali questioni. Recentemente abbiamo partecipato commossi alla dipartita di Raffaella Carrà: quanta energia e quanta voglia di emancipazione c'erano nelle sue canzoni e nei sui balli. È stato rimarcato da molti che per la liberalizzazione dei costumi ha fatto più lei che tanti convegni e trattati. La società, insomma, andava avanti in modo ordinato, ma deciso e lo faceva senza la necessità di leggi e leggine inutili o addirittura dannose. La politica, una certa politica, con la proposta che oggi stiamo discutendo ha fatto sensibili passi indietro. I cambiamenti nel costume e nella società avvengono quando sono percepiti come tali dalla cultura del tempo e non certo per un'imposizione normativa. La proposta in oggetto in questo senso segna un deciso arretramento, tanto nel metodo, per come appena detto, quanto nel merito. Le riserve che si possono muovere al disegno di legge Zan nel merito sono molteplici. Il provvedimento è normativamente inadeguato, giuridicamente pericoloso e politicamente avulso dal sentire dei tempi. Sotto il profilo normativo, le leggi del codice penale che hanno tutelato l'integrità fisica, punendo l'omicidio, le lesioni personali e la violenza privata, al pari di quelle che tutelano la dimensione morale, censurando la diffamazione, l'ingiuria e la calunnia sono pienamente già in vigore e non distinguono il sesso o il genere della vittima; obbediscono coerentemente al principio di uguaglianza dei cittadini sancito nell'articolo 3 della Costituzione. Se l'intento della legge fosse stato quello di tutelare le vittime di discriminazioni sessuali, sarebbe stato sufficiente aggiungere tale necessità alla cosiddetta legge Mancino. Questa aggiunta avrebbe trovato ampio consenso in Parlamento e semplificato l'*iter* della sua approvazione. Il sospetto è che, però, persegua finalità ideologiche, nemmeno molto velate, quelle cioè di normare l'ideologia genderista, che è il più potente movimento di pensiero creato dall'Occidente negli ultimi trent'anni. Sotto il profilo giuridico, si sottolineano tre dati. In primo luogo, le definizioni artificiose dell'articolo 1, che distingue tra sesso, genere, genere, orientamento sessuale e identità di genere, che sembra una costruzione di pensiero che risponde a una ideologia predefinita piuttosto che a una reale esigenza sociale o giuridica.

e così tutto e il contrario di tutto potrebbe essere ritenuto da un giudice propaganda, con buona pace della tassatività quale principio ispiratore di ogni fattispecie penale. In terzo luogo, c'è l'articolo 4 del disegno di legge Zan, che introduce la cosiddetta clausola salva idee: a tal proposito viene in mente, per associazione di idee, un famoso detto latino *excusatio non petita, accusatio manifesta*. In pratica la norma - consapevolmente o no poco importa - mette a nudo i suoi stessi limiti. Se così non fosse, qual era la necessità di inserire questa disposizione? In sintesi, l'approvazione del provvedimento in esame è inutile, anzi, è giuridicamente pericolosa, proprio perché mette a rischio le più elementari e imprescindibili libertà fondamentali da sempre riconosciute e tutelate dalla Costituzione e dall'ordinamento giuridico italiano. I limiti della disposizione sono insomma giuridici e politici. Relativamente a quest'ultimo profilo si mette in evidenza come i costumi non hanno bisogno di prescrizioni normate; si affermano nella coscienza civile e diventano prassi consolidate e nel tempo, quando è necessario, anche disposizioni di legge. Si vorrebbe imporre un elemento che - si ribadisce - ha un fondamento ideologico ben definito, ma tutt'altro che condivisibile e non ci sembra che lo scopo della politica sia questo; anzi, ritengo che dovrebbe essere tutt'altro. Peraltro, non può non osservarsi un forte sostegno a questo disegno di legge da parte di molti personaggi estranei alla politica e il sostegno è stato dato facendo leva su una comunicazione emotiva; è stata ammantata da *cliché* strani dal tessuto civile del Paese; un'operazione di non verità di cui proprio non si sentiva il bisogno. Noti *influencer* amati dai giovani sono scesi in campo per sostenere questa legge. Naturalmente sono liberissimi di farlo, ma c'è da chiedersi il perché e quali siano gli obiettivi di tale campagna. Una cosa, però, è certa: come si conviene a una comunicazione rapida, non c'è approfondimento nei contenuti, ma un orchestrato sensazionalismo dal quale la politica dovrebbe prendere le distanze, anziché fare leva per raggiungere i propri obiettivi. Detto ciò, le parole di questi *influencer* vengono ascoltate da tutti con attenzione, anche da chi ha opinioni differenti, come me, ma mi piacerebbe che anche le parole della Santa Sede venissero ascoltate con analoga attenzione, se non altro perché incarna oltre duemila anni di storia e, quindi, le sue idee vanno ben oltre le contingenze dei tempi. Invece, non è così: si guarda alla Santa Sede con un'ipocrita condivisione quando le posizioni coincidono con i sedicenti progressisti e improvvisamente la stessa istituzione torna a essere oscurantista quando esprime opinioni e idee differenti dalle loro.

Per inciso, la Santa Sede ha voluto porre formalmente all'attenzione del Governo il problema della libertà religiosa, della libertà educativa, della libertà di opinione.

vengono bocciati senza appello. Presidente, per Giacomo Leopardi nessuna qualità umana è più intollerabile dell'intolleranza

definizione limpida di un percorso giuridicamente molto chiaro e netto all'esito delle autorevoli audizioni che si stavano susseguendo. Dispiace poi per il cambio che vi è stato per arrivare alla discussione in Aula perché il disegno di legge in esame, lungi dall'essere uno strumento di tutela contro le discriminazioni, costituisce un pericoloso strumento di limitazione della manifestazione del pensiero in materia di sessualità, volendo di fatto imporre una visione antropologica alla base della teoria *gender*, che nega la dimensione sessuale dell'individuo. Quanto appena si ricava dal fatto che il disegno di legge è formulato attorno a un concetto controverso di identità di genere, elemento alla base della teoria *gender*, al quale i promotori hanno più volte ribadito di non voler rinunciare, malgrado diverse criticità emerse anche nel confronto limitato in Commissione e ora pure in Aula e messe in evidenza anche da autorevole dottrina. gli stessi sostenitori del disegno di legge n. 2005 ci sono state posizioni piuttosto critiche circa il riferimento all'identità di genere, termine considerato vago

e sufficiente determinatezza alla base del nostro attuale ordinamento penale. È quindi plausibile ritenere che la genericità delle norme e la previsione della sanzione penale in caso di violazione determinerebbero come effetto quello di indurre le persone a evitare di manifestare in pubblico il proprio pensiero sul tema della sessualità e su tutte le questioni a esso relative. Si tratta di questioni come, ad esempio, l'adozione da parte di coppie omosessuali, la maternità surrogata o l'educazione dei minori nelle scuole, che necessitano - invece - di un confronto rispettoso e aperto, a tutela della società e delle sue componenti, soprattutto più giovani, per evitare che, in assenza di un dibattito, si radichino concezioni prive di fondamento scientifico e si impedisca la possibilità di aderire legittimamente a visioni della vita e dei rapporti diverse da quelle che si vorrebbe imporre attraverso l'esclusione del dialogo. Pertanto, per la vaghezza dei termini e per il ricorso allo strumento della sanzione penale, in questo caso inadeguato, il disegno di legge pone in serio pericolo la libertà di manifestazione del pensiero e, favorendo l'imposizione di fatto di un pensiero unico, si pone altresì in contrasto con il fondamentale principio pluralistico che costituisce l'architrave del carattere democratico del nostro ordinamento. Due presupposti posti alla base dello stesso - l'emergenza sociale e il presunto vuoto normativo appaiono privi di fondamento. Gli stessi dati forniti dall'Oscad, l'osservatorio del Ministero dell'interno, dimostrano in maniera palese come l'argomento dell'emergenza sociale appaia strumentale, in quanto le stesse segnalazioni relative ai crimini di odio pervenute negli ultimi riguardano principalmente razza, etnia e religione e soltanto in minima percentuale l'orientamento sessuale, il che esclude che si possa parlare di un'emergenza sociale così come viene narrata. Dalla mera lettura del codice penale e dall'esame della giurisprudenza che si è susseguita nel corso degli anni circa i reati commessi in relazione all'orientamento sessuale delle vittime, risulta evidente che non vi sono neppure dei vuoti normativi rispetto a un quadro ordinamentale molto chiaro e compiuto. Nel nostro ordinamento sono già sanzionate le offese, le percosse e le violenze commesse ai danni di chiunque, di qualunque persona senza alcuna distinzione. Lo stesso codice penale prevede anche alcune aggravanti, come la minorata difesa e i motivi abietti e futili, che in ogni caso trovano applicazione anche nei casi di reati commessi in relazione all'orientamento sessuale della vittima. Il disegno di legge in esame, per come formulato, esclude o comunque ostacola il pubblico e legittimo confronto sociale sulle tematiche relative alla sessualità, pretendendo di imporre un pensiero dominante. Quanto detto porta a ritenere che, laddove il disegno di legge venisse approvato, vi sarebbero comunque delle ripercussioni e dei riflessi importanti in quanto la limitazione della libertà di manifestazione del pensiero potrebbe riguardare tutti gli ambiti in cui si svolge la vita sociale. L'ambito maggiormente colpito, come appare poi dal prosieguo la scuola, ove la compressione della libertà di manifestazione del pensiero potrebbe produrre effetti negativi in tema di limitazione di libertà educativa dei genitori che, nel manifestare contrarietà a certi insegnamenti o attività, potrebbero essere ritenuti colpevoli. Limitazione della libertà di insegnamento: gli stessi insegnanti che manifestassero opinioni contrarie potrebbero essere accusati di discriminazione, anche con conseguenze sul piano strettamente e squisitamente professionale, oltreché giuridico. Grave pregiudizio per la formazione scolastica dei minori, che sarebbero privati di un ambiente aperto e pluralista, con una compressione delle capacità di critica e confronto di opinioni. Lo stesso interesse a diffondere la cultura *gender* nelle scuole è stato manifestato chiaramente in vari dibattiti anche pubblici e si evince nitidamente dall'articolo 7, comma 3, dello stesso che prevede il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 dello stesso articolo, ossia per la promozione della cultura del rispetto e dell'inclusione unicamente basata, però, sul tema dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. prevede quindi l'istituzione della Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, finalizzata alla promozione della cultura del rispetto e dell'inclusione limitatamente all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Le scuole di ogni ordine e grado, secondo quanto previsto dal combinato disposto dei commi del predetto articolo, sono chiamate ad organizzare cerimonie e incontri ed ogni altra iniziativa utile per la realizzazione delle presunte finalità. finalità. È singolare riscontrare, in un disegno di legge che formalmente intende introdurre misure di prevenzione e contrasto della discriminazione per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale e sulla disabilità, una palese mancanza di attenzione verso una categoria che pretenderebbe di tutelare: non si comprende infatti per quale ragione la disabilità sia stata esclusa da questa giornata nazionale *(Applausi)* e dalle relative cerimonie e attività previste al comma 3 dell'articolo 7. Di certo la ragione non può rinvenirsi nel fatto che esiste già una Giornata internazionale delle persone con disabilità, posto che esiste già anche la Giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia. A ben vedere, detta esclusione è del tutto priva di fondamento e di valide motivazioni, e sembra piuttosto dovuta al fatto di voler concentrare l'attenzione unicamente sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. legge in discussione possa essere modificato e si possa trovare una sintesi, che abbiamo fortemente portato avanti. Eravamo ad un passo dal raggiungimento di un accordo su piccoli ed elementari accorgimenti: uno per tutti l'articolo 1, quando si poteva passare dalle definizioni finalmente alle finalità. Era questo uno snodo essenziale su cui sembrava raggiunta una convergenza, ma purtroppo andata in un altro modo; mi auguro che il prosieguo possa essere d'ausilio anche alla riflessione rispetto alle notazioni che non sono state portate avanti in maniera compiuta in Commissione giustizia ma dall'esame ampio che sta avvenendo in Aula, si stanno ben rappresentando. Presidente, nella scorsa legislatura sono stato mediaticamente massacrato per aver espresso molti dubbi sulla norma riferita all'adozione da parte di coppie dello dello stesso sesso. Li avevo espressi, continuo a farlo e chiedo rispetto per le mie idee diverse; non faccio riferimento al mio Gruppo parlamentare, che ha sempre rispettato il mio pensiero. Signor Presidente, con riferimento al disegno di legge non c'è da nessuna parte, nemmeno minimamente, un attacco al concetto di famiglia uomo-donna, eppure in quest'Aula l'ho sentito; non c'è da nessuna parte riferimento alle adozioni, all'utero in affitto, eppure in quest'Aula l'ho sentito. Nonostante ciò, si utilizza strumentalmente questo disegno di legge per creare spartiacque elettorali; si droga l'opinione pubblica spacciando menzogne. Veniamo al disegno di legge. La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, nell'uguagliare tutti i consociati indipendentemente dalle diversità di posizione economica, culturale e sociale, introduce l'idea universalistica di un nocciolo di diritti propri di ciascun individuo. Tutti gli individui venivano sottoposti alla medesima regolamentazione racchiusa nella legge. Tale Dichiarazione ha segnato l'evoluzione costituzionale successiva delle Carte flessibili e di quelle rigide, come la nostra. L'uguaglianza, infatti, quale principio indefettibile, viene sancita dall'articolo 3 della nostra Carta fondamentale in un'accezione formale al comma 1 e in una accezione sostanziale al comma 2. Fra i due commi dell'articolo 3 della nostra Carta, non si verifica alcuna contrapposizione logica. La Corte costituzionale ha infatti rilevato che il secondo comma dello stesso articolo 3 della Costituzione - oltre a stabilire un autonomo principio di uguaglianza "sostanziale" e di parità di opportunità tra tutti i cittadini nella nella vita sociale, economica e politica - esprime un criterio interpretativo che si riflette anche sulla latitudine e sull'attuazione da dare al principio di uguaglianza "formale", nel senso che ne qualifica la garanzia in relazione ai risultati effettivi prodotti o producibili nei concreti rapporti della vita, grazie al primario imperativo costituzionale di rimuovere i limiti "di fatto" all'uguaglianza e di perseguire l'obiettivo finale della "piena" autodeterminazione della persona e partecipazione alla vita comunitaria». Il principio di uguaglianza è strettamente collegato al divieto di distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali.

«oppure fondati (...) sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere» si pongono nel solco dell'evoluzione del principio di uguaglianza.

aggiungendo ad alcune delle condotte ivi richiamate i motivi di discriminazione fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità. Capiamoci meglio: attualmente l'articolo 604-*bis* del codice penale punisce «chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi», o chi commette «violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi». A tutto questo, pertanto, si aggiungerebbe semplicemente «oppure fondati (...) sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere». Ce lo vogliamo dire o non ce lo vogliamo dire che esiste un problema che vede ancora tante persone, che hanno condotte anche molto violente, fondate sulla discriminazione di sesso, di genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità, oppure facciamo finta di nulla? A questo punto finisco con alcune osservazioni specifiche, un po' più tecniche, anche sostanziali, e mi faccio aiutare da un messaggio che mi è pervenuto da un'amica, che chiamo Monica, sposata con dei bambini, a cui piace anche molto il marito: «Caro Sergio, ormai sono molti anni che sei senatore e io (ma vedo che siamo un po' tutti sulla stessa linea tra amici) ho cercato, per quanto possibile, di evitare le discussioni su temi caldi del momento in politica, salvo magari qualche discorso di ordine generale. Questo non tanto perché temevo di dare l'impressione di voler spingere su questioni personali (è tutto su un piano di tale integrità che il dubbio non sfiora nemmeno nessuno di noi), ma perché pensavo fosse giusto lasciarti respirare e pensare ad altro, nel momento in cui eri tra amici. Questo per farti capire quanto ho dibattuto con me stessa prima di mandarti queste righe. Da madre e da insegnante il dibattito su questo ddl Zan mi ha estremamente coinvolto in questi mesi e purtroppo ora vedo che c'è un rischio concreto che questa legge non passi al Senato, forse per pochi voti. So che il MoVimento 5 Stelle sarebbe propenso a votare a favore, ma certamente avrete contatti anche con indecisi o con senatori che intendono votare contro. Io vi porto la mia esperienza, per quel che vale, e puoi comunicarla a chi vuoi con il mio nome e cognome»; va bene Monica. «Ieri mia figlia, di ritorno da un campo estivo della parrocchia, che ironicamente ha proprio come tema il rispetto delle diversità, mi ha raccontato che un ragazzino di quattordici anni è stato allontanato per aver offeso uno degli animatori con l'epiteto di "ricchione". Nella mia classe una ragazzina di dodici anni ha confidato quest'anno a noi docenti di aver avuto sempre dubbi sulla sua identità di genere, in quanto non si riconosce nel genere femminile. Ne abbiamo parlato con molta serenità sia con lei che con la famiglia, per fortuna molto accogliente. Ecco un chiaro caso in cui si applica l'articolo 1 del disegno di legge. Come potrebbe una ragazzina di dodici anni aver completato un percorso di transizione? È naturale che in questo momento il genere per lei sia solo un qualcosa di percepito; un domani con calma si vedrà, ma se questa ragazzina oggi fosse fatto oggetto di discriminazione e di violenza, perché si percepisce maschio, vogliamo lasciarla senza tutele solo perché il suo percorso di transizione non è, né potrebbe essere ancora iniziato? Io sono molto meravigliata e addolorata dal fatto che si utilizzino i drammi di bambini e adolescenti emarginati per la loro diversità per fare politica» - me l'ha scritto appositamente con la "p" minuscola «per alleanze e consensi. Ancor di più, da cattolica, sono basita dalla continua paura mostrata nei confronti di una legge a tutela di una parte debole. Veniamo ora all'articolo 7. Vi posso assicurare che a scuola ogni anno siamo inondati di ricorrenze, di giornate di ricordo "x" e contro "y". In tutti questi casi, celebrare la giornata e come effettivamente farlo scelta del singolo istituto, tramite i suoi organi collegiali (collegio dei docenti e consiglio d'istituto). Perciò si fanno delle scelte, anche perché, se volessimo partecipare a tutto, non avremmo più tempo di fare lezione. Questa paura dell'indottrinamento obbligatorio è del tutto infondata e inoltre al massimo la scuola potrebbe liberamente scegliere di limitarsi a un richiamo al rispetto del prossimo e a evitare delle discriminazioni, cosa che ogni scuola di un Paese civile non può che desiderare di trasmettere ai suoi allievi. disegno di legge al piano dell'offerta formativa triennale e al patto di corresponsabilità tra scuola, studenti e famiglie assicura già da solo e a sufficienza che tutti gli attori coinvolti siano informati e d'accordo; anzi, è pure pleonastico secondo me. C'è ovunque un eccesso di cautela in questo disegno di legge, come se le paure di persone e organizzazioni fossero più da tutelare che non le minoranze stesse che la legge intende tutelare. Ma sono loro in pericolo, non l'opinione pubblica. Non è la prima volta che un adolescente *gay* mi confida di doversi appartare in luoghi il più possibile isolati per scambiarsi un bacetto, cosa che noi appunto» sto concludendo, Presidente - «raccomandiamo costantemente ai nostri figli di non fare, per la loro sicurezza. Concludo ricordando che ogni professore, genitore di ragazzo LGBT, educatore parrocchiale potrà riportarvi infiniti episodi di omo-, lesbo-, bi-, bi-, transfobia di cui sono vittime dei minorenni. Ti ringrazio di aver seguito queste mie lunghe riflessioni e ti invito nuovamente a farne l'uso che ritieni più opportuno». Eccolo, Monica, a presto. *(Applausi)*.

sono contenta che Fratelli d'Italia abbia deciso questa maratona contro questa proposta di legge, perché, vedete, questa proposta di legge non è contro le violenze, contro le discriminazioni e a favore degli omosessuali. Credo che in tutta quest'Aula sarebbero tutti d'accordo, compresi noi di Fratelli d'Italia, se parlassimo di discriminazioni o di atti di violenza contro gli omosessuali. Vi ricordo che la scorsa settimana

anzi, meglio se lo si riesce a mettere in carcere. E non vorrei che qualche collega mi rispondesse che questo non è possibile. Vi voglio citare degli esempi accaduti in altri Paesi, dove abbiamo leggi simili a quella che voi volete approvare. È successo a un cardinale, ad esempio, che è stato indagato per aver detto che la famiglia è formata da un uomo e da una donna. È successo a un padre di famiglia, che ha passato una notte in carcere semplicemente perché, andando a una manifestazione *prolife*, aveva una maglietta bianca con scritto «Viva la famiglia». Quindi non veniteci a dire, come sentiamo in molti interventi, che non è vero che questo disegno di legge vuole tappare la bocca a chi è contro

volete cancellare tutto. Tutto deve essere fluido, non c'è più l'appartenenza di genere, non ci sono più le nostre radici, non c'è più niente. Dobbiamo diventare esseri fluidi. Questo è il modello che volete imporre e al quale invece noi, con tutte le nostre forze, ci ribelliamo. È il politicamente corretto,

dalla mattina alla sera. *(Applausi)*. Non è consentito che qualcuno non la pensi alla vostra maniera e questo è gravissimo. Noi stiamo subendo, sì, violenza, odio e discriminazione, perché nessuno di noi

invece, in questa proposta di legge, si parla di odio, che è la cosa più grave. Si parla di discriminazione, ma per il proprio pensiero. proprio pensiero. Colleghi, fate un'altra riflessione. Vi sembra giusto, su una materia così complicata, delicata e difficile, anche nella sua spiegazione, lasciare tanta discrezione ai magistrati? Io sono terrorizzata. Ci sono tantissimi magistrati in Italia che fanno assolutamente bene il loro lavoro, con passione, con dedizione e con equità. Ma abbiamo una piccola parte di magistrati che sono ideologicamente e politicamente esposti. E io domani devo essere giudicata da uno di questi, che magari nel suo giudizio impone la sua ideologia, che è uguale al vostro modello? Io credo che tutto questo dovrebbe preoccuparci. Una cosa che mi preoccupa profondamente è che lo Stato di diritto lo Stato di diritto dovrebbe occuparsi dei più deboli, di coloro che non hanno possibilità di difendersi, ossia dei bambini. I bambini sono completamente dimenticati

farlo gli omosessuali. È vero che la vita impone e ha imposto ad alcuni di noi di non avere, magari, il padre e la madre, ma non per una legge dello Stato, che decide, per legge, che un bambino possa fare a meno del padre o della madre. Ma vi rendete conto di quello che state portando avanti, del modello che volete imporre? Mi rivolgo poi a molte donne, alcune femministe, che hanno combattuto per i diritti delle donne. Ma vi sembra giusto - faccio un esempio finanche un po' banale, ma che è sotto gli occhi di tutti e che sta già avvenendo - che nelle competizioni sportive

la discriminazione e la violenza. Per noi di Fratelli d'Italia ci sarebbe un modo per combatterle, ed è una proposta che ha avanzato che ha avanzato Giorgia Meloni. Come mai l'Italia, e nessuno di voi (lo dico a tutti) ha mai detto una parola sul fatto che abbiamo rapporti commerciali con Paesi dove dove l'omosessualità è un reato e dove si punisce financo con la pena di morte, come il Qatar, dove ci saranno i mondiali, come l'Arabia Saudita? E come mai non vi stracciate le vesti quando un omosessuale può essere addirittura punito con la pena di morte? Non vi fa sobbalzare sulle vostre sedie? Non fa aprire un dibattito, se veramente tutti ci tenessimo a difendere gli omosessuali dalle violenze e dalle discriminazioni? Gli omosessuali, quelli orgogliosi, non si fanno strumentalizzare né dalle *lobby gay*, né da voi.

userà tutti gli strumenti a disposizione del nostro sistema per combattere, perché credo che se dovesse passare questo disegno di legge, verrebbe imposto un modello che è il contrario di quello che noi vogliamo per il futuro dei nostri figli.

parto col dire chiaramente che sono e sarò sempre contro ogni violenza e ogni discriminazione per motivi di sesso, di genere, di identità sessuale e di orientamento. La mia storia, anche parlamentare, lo può testimoniare e per quanti ci ascoltano magari da casa questo va detto, perché nel dibattito che ho ascoltato in questi giorni, settimane, mesi (come se non fosse in atto una crisi economica e sociale gravissima), sembra che tutto si limiti a classificare, talvolta anche con arroganza e spesso con pregiudizio, chi è a favore e chi è contrario al disegno di legge che stiamo discutendo. Chi critica il disegno di legge al nostro esame è attaccato come omofobo, senza possibilità di ragionamento. Questa è una strumentalizzazione, e già questo fa venire i brividi, perché sembra che, in luogo di questi valori, cioè in sintesi del rispetto che deve essere valore di tutti, di tutti, ci si arroghi il diritto e la prosopopea di essere gli unici detentori di una verità e del bene comune. Credo piuttosto che in un dibattito così delicato, così importante, etico, valoriale e sociale, i toni che si dovrebbero utilizzare dovrebbero essere certamente più pacati, pieni di responsabilità, consapevolezza, coscienza di quello di cui si sta parlando. Il problema di questo disegno di legge è il più grande ed evidente che hanno tutte le leggi scritte male, piene di commi e rimandi normativi. Io Io sono un medico, non sono una giurista, è vero, ma ho imparato negli anni la prima regola fondamentale della buona scrittura delle leggi. Il tema della buona scrittura delle leggi rappresenta un aspetto della più generale questione della qualità della legislazione, che a partire dagli anni Ottanta si è imposta all'attenzione del legislatore. Si è rilevato in particolare come l'ipertrofia normativa, con il proliferare di regole e prescrizioni a carico dei cittadini, famiglie (non so fino a quando si potrà dire questa parola) e imprese, ed il diffuso stato di incertezza normativa, dovuto a carenze nella qualità della legislazione, in termini sia formali sia sostanziali, abbiano prodotto e producano un costo oltre che per l'economia, per la democrazia, in quanto riducono l'effettiva conoscibilità dell'ordinamento giuridico da parte di coloro che vi sono soggetti. Dunque, credo che il disegno di legge al nostro esame pecchi proprio in questo: lascia ai magistrati e alla magistratura ampio spazio di interpretazione. Non è la magistratura ad arrogarsi questo diritto, è il legislatore che, come spesso accade, depone la sua funzione, non si assume la piena responsabilità e lascia invece alla magistratura ampio spazio e il dovere di decidere. Come anche lascia i cittadini nella condizione di doversi dimenare da soli se un'opinione e l'espressione di essa sia un reato perseguibile penalmente oppure no. Tant'è che gli interrogativi che vengono alla mente sono tanti. Sarà reato, ad esempio, riconoscere la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio? Sarà reato dire che il matrimonio è una unione tra un uomo e una donna? Sarà reato dire che è inaccettabile generare attraverso l'utero in affitto, perché è una barbarie usare il corpo della donna come fosse un'incubatrice meccanica? Sarà reato accettare un uomo che si sente donna in una squadra di calcio femminile? Sarà reato non inserire nelle quote rosa un uomo che si sente una donna? Cito il caso di un conoscente, un amico di mia figlia, che, per farsi assumere per uno *stage* presso una grande banca di investimenti a Londra, una multinazionale che riserva, appunto, quote per i *gay*, si è finto *gay*, approfittando delle quote loro destinate. Questa è la vera mancanza di rispetto. Questa è la mancanza dei diritti. Il caos che si genererà, se questa legge verrà approvata senza modifiche, sarà questo. Queste domande qualcuno le ha poste a se stesso? Il furore ideologico che si cela dietro il disegno di legge Zan, confermato dall'insindacabile fermezza con la quale una parte politica dice che no, deve essere approvato così, non si ferma davanti a niente, nemmeno davanti ai bambini, che andrebbero lasciati fuori dal dibattito politico. Ai bambini si deve insegnare il rispetto per tutti, per gli esseri umani, per gli animali, per la natura, perché, rispettando gli altri, rispettiamo noi stessi, nonché il rispetto per i nostri valori e le nostre idee. I bambini non devono essere strumentalizzati come è stato fatto per sostenere l'approvazione di un disegno di legge. Noi dobbiamo insegnare a rispettare le diversità, perché ognuno di noi è diverso dagli altri. Ognuno di noi ha il diritto di essere rispettato.

Si toglie alla famiglia, con una legge, la responsabilità educativa, soprattutto in temi così delicati, la cui conoscenza dipende dal grado di maturità di ogni bambino. Il fatto che a Bologna, in occasione del *Gay Pride*, gli organizzatori abbiano sfilato indossando una mitra vescovile, calpestando con vernice rossa i volti di vari personaggi, tra cui anche il Papa, secondo voi non è palesemente lesivo dei principi democratici necessari per organizzare una manifestazione pubblica, che non fa altro che promuovere odio verso i cattolici e i politici che si sono schierati contro questo disegno di legge? Mentre l'Italia e l'Europa vivono una vera emergenza legata al calo della natalità e all'inverno demografico, "L'Espresso" ha pubblicato una copertina a mio avviso inappropriata, se si può dire ancora, per la Giornata internazionale contro omofobia. Potrò continuare a sostenere che mi oppongo fermamente al concetto di uomo incinto o sarò accusata di omofobia? Non la forza, ma la costanza di un alto sentimento, fa gli uomini superiori. Ricordatelo. Cosa accadrebbe se il disegno di legge Zan fosse approvato al Senato così com'è, senza modifiche? Piccole richieste, sostanziali, e la legge sarebbe approvata in una settimana, come è stato detto da vari esponente del centrodestra. Ora, tra le polemiche dei sostenitori, che non so elencare, visto che hanno avuto a mio avviso anche fin troppa visibilità, abbiamo avuto una prova molto concreta. È accaduto che Antonio Tajani, vice presidente di Forza Italia, ha detto che la famiglia per noi è il nucleo fondamentale della società, che va difesa le nostre politiche sono sempre state a sostegno della maternità. Ad esempio, nel *recovery plan* presentato dal Governo italiano a Bruxelles, c'è una parte consistente sugli asili nido. Noi continuiamo e continueremo ad andare in quella direzione. Ora, vi sembra di aver ascoltato in questa dichiarazione un qualche attacco omofobo, una discriminazione, un'intolleranza, un'offesa alla comunità LGBT, una riduzione dei diritti delle libertà di *gay*, lesbiche e *transgender*? A me non sembra. Eppure si è gridato subito allo scandalo e al reato d'opinione e ne è scaturito un diluvio di attacchi, solo per aver ricordato che la famiglia è un nucleo fondamentale della società e che va difesa. La famiglia: quella che evidentemente tutti vogliono che muoia, portando via con sé la cultura, l'arte e le tradizioni del nostro Paese. Volete dissolvere il più forte istituto sociale. Le famiglie italiane sono circa 25 milioni. Ho sentito dire in quest'Aula che siamo nel 2021, come se il rispetto dell'essere umano dovesse avere una temporalità: vale nel 2021, varrà tra cinque anni ed era insegnato cinque anni fa. Credete che basti una legge farraginosa per impedire di insultare qualcuno? Ne abbiamo la prova, perché altrimenti le carceri sarebbero vuote. disegno di legge scritto male, che rende più ambigue situazioni che non necessitano di ambiguità, difende i diritti di alcuni, attaccando quelli degli altri. È questo il suo scopo? È questo che volete insegnare? A questo disegno di legge, così com'è, dico no. *(Applausi)*.

colleghe e colleghi, prima di entrare nel merito del provvedimento in esame voglio lasciare all'Assemblea delle riflessioni sul Presidente della Commissione giustizia, il senatore Andrea Ostellari, anche, ma non soltanto, alla luce dei rilievi ingiusti che nell'ultima seduta sono stati mossi nei suoi confronti. Intanto voglio esprimere - sono convinto di poterlo fare in nome e per conto di gran parte dell'Assemblea - la solidarietà nei confronti del Presidente, per gli attacchi ingenerosi, strumentali ed infondati che ha ricevuto. Allo stesso tempo, nei suoi confronti voglio esprimere apprezzamento per il modo in cui ha condotto il suo ruolo di Presidente, soprattutto nella gestione di questo affare. Esprimo questo apprezzamento

per lo sforzo enorme che ha profuso per addivenire ad un accordo, che poi è stato portato avanti dal nostro capogruppo Romeo e, fino a poche ore fa, dal nostro capo politico, Matteo Salvini, voglio esprimere nei confronti del presidente Ostellari profonda ammirazione, perché ha messo in campo un'azione politica, che era anche al di là del ruolo istituzionale che ricopre. La politica, quella sana e buona, normalmente tende ad unire e ancor di più bisognerebbe unire, quando si tratta, come accade in questo caso, di diritti. Un Paese e un'istituzione si uniscono, non si dividono. del Partito Democratico, di Liberi e Uguali e del Movimento 5 Stelle, avete diviso tutto ciò che si poteva dividere. Alla fine, avete diviso anche l'atomo e avete diviso il Paese.

i mal di pancia nel Partito Democratico ormai sono noti, così come sono noti i mal di pancia all'interno del MoVimento 5 Stelle. Avete proposto, secondo il vostro punto di vista, una rivoluzione in termini di diritti civili e vi siete messi finanche nelle mani di Ciampolillo. Volete fare una rivoluzione nel Paese, ma avete respinto una questione sospensiva grazie al ritardatario Ciampolillo: diciamo che i presupposti per una rivoluzione non ci sono, né nel contenuto, né tantomeno

ci si aspetta che venga indicato il viatico verso una soluzione unitaria, di buon senso, matura. Invece no, c'era tanta acredine. È vero, allora, quanto si dice: predicate amore, ma diffondete odio. Questo non va assolutamente bene. Fermatevi, Fermatevi, scendete con i piedi per terra e cerchiamo di offrire a centinaia di migliaia di persone una legge utile, aderente aderente alle loro aspirazioni, ai loro bisogni. Se qualcuno mi dovesse chiedere se siamo favorevoli a una legge contro le discriminazioni nei confronti di omosessuali, transessuali, lesbiche o persone di qualsiasi orientamento sessuale, risponderei di Se qualcuno invece ci dovesse chiedere se siamo favorevoli a una legge contro la libertà di pensiero, che porti la teoria gender nelle scuole, che invada la vita dei bambini, che addirittura parli di identità di genere, direi di Quel sì e quel no sono perfettamente compatibili, perché una legge che limita la libertà di manifestazione del pensiero e che invade la vita dei bambini non ha nulla a che vedere con la tutela contro le discriminazioni di qualsiasi tipo. *(Applausi)*. Qual è la soluzione? Togliamo da questa dialettica, non permettiamo che venga estesa la legge Mancino e che quindi ci siano ulteriori restrizioni nei confronti della libertà di manifestazione del pensiero; sgomberiamo il campo dalle ideologie e dalle bandierine - oserei dire dai marchi politici che a tutti i costi cercate di imprimere - e mettiamo al centro i diritti. Il diritto di amare chiunque; è stato detto: siamo tutti quanti ultra favorevoli; il diritto di opinione, il diritto di crescere serenamente. I bambini non devono essere asfissiati da questa vostra volontà; devono poter giocare e sognare e, nel momento in cui diventeranno adulti, decideranno della loro vita. il diritto dei genitori - che diventa anche un dovere - di educare i loro figli secondo l'indirizzo familiare, e questo non lo diciamo noi; lo dice la Costituzione, all'articolo 30 recita: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli». Lo dice l'articolo 2 del protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: «Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche». Non potete scippare ai genitori questo diritto che diventa anche un dovere. Eliminate i capricci, parliamo di diritti. Togliete i capricci perché il fatto di poter avere un'identità, una percezione a piacimento, è un capriccio, non riguarda un diritto. E ritorno a quanto aveva proposto il presidente Ostellari: c'era e c'è ancora la possibilità - auspichiamo fino all'ultimo che si concretizzi - di mettere in campo una legge di civiltà, una legge di buon senso. Abbiamo affrontato l'articolo 1 (via l'identità di genere), l'articolo 7 (via la teoria gender dalle scuole) parliamo dell'articolo 4, ma questo è un costume un po' grillino: individuare una fattispecie penale vaga, indeterminata. Ricorderete qualcuno alla Camera dei deputati che aveva sostenuto la teoria della vaghezza della norma penale, mentre deve essere l'esatto contrario, perché la norma penale deve essere chiara, puntuale e precisa, per un semplice e banale motivo: perché quando ci si sveglia la mattina si deve sapere ciò che è lecito e ciò che non lo è, e l'articolo 4 di questo testo non lo permette. Si può lavorare con l'inasprimento delle pene per le fattispecie già previste; è stato proposto un ampliamento dello spettro di fattispecie che possono integrare violazioni, violenze, discriminazioni da avversare e si può lavorare su questo versante.

Il più grande responsabile è il segretario del Partito Democratico, che innanzitutto non sta avendo rispetto di questo Parlamento; non sta avendo considerazione delle varie sensibilità che con tante argomentazioni sono emerse. Ma soprattutto, non ha rispetto di questa istituzione, visto che si appresta a farne parte, salvo che decida di prendere la via della Tour Eiffel, dove magari potrà tornare a fare ciò che ha fatto prima e che lo ha fatto di gran lunga peggiorare. un'ultima considerazione. La scorsa settimana - lo dico con rispetto, ma con fermezza - ho visto diverse mascherine arcobaleno tra tra questi banchi, adesso non ne vedo più nemmeno una e non so se significhi qualcosa. Addirittura vedo i banchi vuoti, per cui evidentemente il vostro interesse verso questo disegno di legge va sempre più scemando. Voglio dire, però, che potete indossare 10, 100, 1.000 mascherine, ma se non contribuite a portare a casa una legge buona per queste persone, non avrete reso un buon servizio né al Paese, né a queste persone.

ho sentito dire in quest'Aula che questo disegno di legge non serve, ho sentito dire che abbiamo altri problemi. Ebbene, Presidente, qualcuno provi a dirlo a chi è bullizzato, a chi è discriminato per i propri sentimenti, per la propria natura; qualcuno provi a dirlo a chi è costretto a subire la paura dell'aggressione, del pestaggio ed è impedito a uscire, a vivere liberamente la propria vita, a mostrarsi per come è. Essere discriminati per la mancanza di lavoro è grave allo stesso identico modo che essere discriminati perché si è donne o per il proprio orientamento sessuale o perché si è disabili, perché diritti sociali e diritti civili stanno insieme, perché la nostra vita, la possibilità di realizzarci è più cose insieme, tutte indispensabili: poter studiare, poter lavorare, poter amare. Non vengo da una formazione laica, ma da una formazione personale cattolica e comunista e so che questo provvedimento è importante perché risponde ad una domanda, ad un bisogno sociale, non solo individuale, perché allargare tutele e diritti civili significa sempre allargare tutele e diritti sociali, gli uni e gli altri solo insieme permettono di realizzare pienamente la propria esistenza, il proprio progetto di vita. Qui sta l'urgenza di questa legge, che parla di vite, di esistenze, di quotidianità, di futuro da poter costruire, in particolare per le nuove generazioni che più sentono sulla propria pelle il tema della discriminazione, dell'intolleranza come un peso sulle loro esistenze. Questa legge contrasta discriminazioni e violenze legate a sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità e basterebbe questo titolo a racchiuderne e a farne capire l'importanza. È una legge che amplia le tutele perché quelle che finora esistono nel nostro ordinamento non bastano e vanno vanno nominate e riconosciute le differenze, anche quelle nuove, e vanno tutelate e questo è quello che stiamo facendo con questa legge, nel pieno solco dell'articolo cardine della nostra Costituzione, l'articolo 3 sull'uguaglianza. Questa legge identifica nuove fattispecie di lesione dell'uguaglianza e le contrasta apertamente, perché per sconfiggere un crimine, un sopruso, bisogna parlarne, averne consapevolezza, denunciarlo, non essere indifferenti o far finta di nulla come fa qualcuno in quest'Aula. Dal 2013 sono 1.294 le vittime di episodi di omofobia,

Dal 2013 sono 1.294 le vittime di episodi di omofobia, 186 nell'ultimo anno. Il mese di giugno 2021, appena trascorso, è stato il più omofobo di sempre: 19 episodi, per un totale di 30 vittime, una al giorno, aggressioni a singole persone, a gruppi, a coppie, come quella denunciata ieri da due ragazze, Francesca e Martina, aggredite in spiaggia. Giugno è il mese dei Pride e molti di questi episodi sono avvenuti contro persone che andavano o tornavano dalle manifestazioni. È inoltre sempre più preoccupante che queste aggressioni vigliacche colpiscano vittime sempre più giovani, in alcuni casi adolescenti di dodici

ragazze e ragazzi pestati, coperti da insulti per uno smalto sulle unghie, per il modo di vestire, per una borsa arcobaleno indossata, per un cappellino con la scritta LGBT, per un bacio scambiato, per delle effusioni su una panchina o per una complicità adolescenziale tacciata di omosessualità: frattura al naso, rottura della mandibola, trauma cranico, rottura della mascella, stalkerizzazione sui *social*. C'è un sito, «omofobia.org», che raccoglie quotidianamente ogni dato di questa *escalation* in tutta Italia. cose vanno viste e lette una ad una e, di fronte a questa enormità, vi chiedo che altro stiamo aspettando. Ogni giorno perso è un insulto a tutto il Paese perché, se uno di noi è discriminato, tutti siamo discriminati. provvedimento in esame va approvato al più presto, così come votato dalla Camera, dopo un dibattito che è stato amplissimo, dopo una profonda riscrittura che c'è già stata. stata. Modificarlo nuovamente, ricominciare daccapo l'*iter* parlamentare significherebbe affossarlo e darla vinta alle destre, che questa legge hanno osteggiato e osteggiano, e non lo dico assolutamente con compiacimento, ma con rammarico. Significherebbe darla vinta a chi da sempre, con tutte le proprie forze e con un atteggiamento strumentale e reazionario - si è visto anche nella discussione in quest'Aula ha cercato di affossare questa legge, come dimostrano i 700 emendamenti della Lega. Altro che mediazione. Questo è l'ostruzionismo di chi non vuole questa legge e vuole affossarla per sempre. Eppure basterebbe mettersi per un attimo nei panni di un ragazzo umiliato e offeso e non ci sarebbero dubbi sulla necessità di approvare la legge al più presto e sono convinto che le forze che l'hanno sostenuta e votata alla Camera devono avere la responsabilità politica aperta e chiara di approvarla in via definitiva qui in Senato, senza modifiche ulteriori che ne metterebbero a rischio i contenuti. Al Paese serve infatti una legge di civiltà e questa lo è, mentre togliere il riferimento alle discriminazioni contro l'identità di genere sarebbe un errore enorme, un passo indietro di decenni per la nostra società, perché l'identità di genere, cioè sentirsi e viversi diversi da quello che c'è scritto sulla carta di identità, è un tema gigantesco, che riguarda le soggettività di ognuno, la complessità esistenziale, la propria autodeterminazione e va rispettato. Già nel 2015 la Corte costituzionale ha parlato di diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, che rientra a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona. Per questo l'identità di genere è oramai ovunque nel nostro ordinamento giuridico e in quello internazionale. Togliere questo riferimento significherebbe eliminare la tutela alle persone omosessuali e *transgender* che la Corte costituzionale riconosce già dal 1985; significherebbe tornare indietro di quarant'anni, svuotare di significato questa legge e passare da una buona legge a una legge sbagliata. Signor Presidente, in conclusione voglio dire basta con le falsità su questo testo, che non limita in alcun modo la libertà di espressione, perché nessuno può scambiare la libertà di pensiero o di parola con l'istigazione alla violenza. infatti, è sempre fondata sul rispetto della dignità altrui oppure diventa sopruso, specie in questo tempo dove il *web* amplifica i discorsi d'odio e crea un clima ostile alle minoranze. questa legge non porta nelle scuole alcun indottrinamento *gender*, ma promuove un'educazione volta al rispetto di ogni persona nella sua diversità affettiva e sessuale,

inviato a tutti i parlamentari e a tutti i senatori hanno scritto molte personalità e associazioni cattoliche raccolte nel progetto Gionata. C'è scritto che la giornata del 17 maggio può diventare occasione

afferma: «ogni persona, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, va rispettata nella sua dignità e accolta con rispetto, con la cura di evitare "ogni marchio di ingiusta discriminazione"». Presidente, è ciò che stiamo provando a fare con questa legge perché pregiudizi, stereotipi e discriminazioni possono distruggere una vita e possono minare una democrazia. Noi abbiamo il dovere di evitarlo e contrastarlo; abbiamo il dovere di tutelare la vita di ognuno e la democrazia di tutti. *(Applausi)*.

non utilizzerò tutto il tempo che ho per il mio intervento poiché, considerata la delicatezza e l'importanza della questione oggetto del disegno non vorrei utilizzare molte parole, che potrebbero anche essere strumentalizzate. Mi limiterò, pertanto, a sollevare alcune eccezioni tecniche. Premesso Premesso che il nobile fine che la legge vorrebbe raggiungere non è assolutamente in discussione, il disegno di legge, però, non è condivisibile nella parte in cui si fonda sul presupposto che, alla tutela degli interessi ivi previsti, possa procedersi attraverso lo strumento del diritto penale. Per come è strutturato in tale parte, il disegno di legge Zan, a prescindere da ogni scelta valoriale che ho premesso all'inizio di questo mio intervento, presta il fianco a problemi di legittimità costituzionale, in quanto introdurrebbe, come notoriamente evidenziato in autorevoli sedi, previsioni incriminatrici prive dei requisiti della certezza e della tassatività. Questo è un fenomeno molto grave e pericoloso. Verrebbe messo in discussione anche l'altro principio fondato sull'effettiva offensività della condotta che si intende punire, in quanto sarebbe difficilissimo tracciare un confine netto tra le manifestazioni di pensiero effettivamente deprecabili e lesivi degli interessi che si intendono tutelare e le altre che, al contrario, costituiscono libera manifestazione di pensiero e, come tali, rientranti nei principi fondamentali garantiti e tutelati dalla Carta costituzionale. Infine, come dimostra la comune esperienza oramai sotto gli occhi di tutti, le norme penali già esistenti e astrattamente applicabili - esistono nel codice già delle norme che possono essere applicate alle fattispecie contemplate nel disegno di legge Zan - hanno dimostrato e mostrato tutti i loro limiti sul piano della prevenzione e dell'educazione. Piuttosto, in base a un diverso approccio, gli strumenti idonei alla professione e al contrasto di queste discriminazioni dovrebbero essere fondati su principi di civiltà e processi educativi e culturali che si fondano sul rispetto della persona umana in quanto tale. Cari colleghi,

hanno la presunzione di tutelare determinati diritti inviolabili delle persone, ma che purtroppo, in alcuni casi,

non solo perché nel merito è chiaramente e in modo evidente illiberale e incostituzionale, ma anche per la modalità con cui oggi il Senato se ne sta occupando. È stato un errore aver insistito perché si accelerasse l'*iter* e non solo perché questo è un provvedimento divisivo. Credo che almeno su questo siamo tutti d'accordo: non è il Parlamento diviso su questi contenuti, lo sono gli italiani e quella società civile che in questo momento sta cercando con grande fatica di riprendere in mano le proprie sorti, insieme all'economia del Paese, e di ricostruire. Credo sia evidente a tutti che ciò sarà possibile anche grazie all'ampia maggioranza che si è assunta le proprie responsabilità e ha voluto metterci la faccia per far ripartire il Paese. Cosa c'entra tutto questo? C'entra con il fatto che questa maggioranza ampia è un'occasione per il Paese - io ci credo - ma a condizione che non giochi all'ideologia e a cercare di trovare ciò che divide invece che ciò che unisce,

a fronte di un'urgenza che non c'è, si cerca di legittimare e imporre a questa Camera un'inerzia come mai è stato Su questioni etiche e di libertà non è mai accaduto che si sia imposto a una delle due Camere di non occuparsene e di stare a guardare (o - meglio - è già accaduto, ma durante il regime fascista). E così, ora si vorrebbe che il Senato venisse meno ai propri compiti, avallando ciò che ci viene passato dalla Camera dei deputati. Si parla di diritti e tutele, ma il vero problema è il pensiero unico che si vorrebbe introdurre con questo disegno di legge. Si sostiene che esso tuteli le coppie omosessuali dando nuovi diritti, ma non c'è niente di più falso di più falso e ingannevole, perché qui il tema non è tutelare persone in condizioni di debolezza, che è un dovere da parte di uno Stato laico: in questa norma l'intento etico-educativo diventa ideologia, assumendo un'ulteriore prepotenza nell'eccessiva volontà di definire l'identità sessuale. Di questo il Paese non aveva bisogno, perché il clima di odio - a cui ha accennato anche il collega che ha parlato precedentemente - temo che abbia anche come origine un dibattito assurdo che qualcuno ha voluto montare nel Paese, con la complicità di personaggi famosi.

una società civile seria e la responsabilità da parte di una politica che sappia dare indicazioni coese e condivise. Di questo oggi ha bisogno l'Italia: di un'indicazione chiara e condivisa, non di una divisione come quella che invece sta nascendo all'interno del Parlamento. proponenti purtroppo sanno che il disegno di legge Zan, così com'è impostato, diventa un cavallo di Troia per l'introduzione del pensiero unico, rendendo il nostro - e non lo dico a caso - uno Stato illiberale, cosa che nessuno di noi può accettare. Per queste ragioni, l'introduzione del reato di opinione evoca regimi fascisti e totalitari. Guai a chi continuasse a dire che non è così e a rendere

L'ideologia di genere non mira a difendere le persone, ragazzi o adulti che siano, che vivono in modo problematico un conflitto tra il proprio corpo e la propria psiche, ma a confondere la realtà, facendo in modo che il soggettivo superi l'oggettivo, con l'idea che nessuno è uomo e nessuno è donna, ma siamo tutti in divenire. Anche questo è inaccettabile. *(Applausi)*. Non si può portare un tema che ha, sì, a che fare con problemi, singoli o anche diffusi, che devono essere affrontati con grande responsabilità da chi se ne deve occupare, e di cui la legislazione deve farsi carico, ma che non c'entra nulla con l'idea che invece debba essere reputato reato

che è chiaramente indipendente dal sesso. Il rispetto e il riconoscimento che dobbiamo ad affettività diverse dalla coppia naturale, però, cosa c'entrano con tutto questo? tutto questo? E cosa c'entrano i bambini, che si vorrebbero crescere educandoli a un'assenza di certezze e radici, dimenticando che il diritto a educare spetta alla famiglia? Se si tratta di trovare ulteriori tutele a condizioni particolari, così come ad aggravare qualsiasi condanna a potenziali violenze, fisiche o morali, credo che nessuno di noi farà mancare il proprio sostegno e tutti faremo la nostra parte. Se però la volontà diventa l'introduzione del pensiero unico *gender*, con l'impossibilità di pensare e affermare il ruolo prioritario - questo sì - della famiglia naturale, allora non potremo che opporci, per amore della realtà e della libertà.

che di tutto hanno bisogno meno che di essere messe al centro di un clima che il nostro Paese sinceramente non dovrebbe vivere. Dovrebbe stare a cuore a tutti approvare una norma che possa dirsi largamente condivisa dal Parlamento, così come dagli italiani.

purché vengano rispettate le leggi. Siamo per il rispetto della libertà di scegliere come vivere il proprio privato. Noi siamo per rigettare, cari colleghi, e condannare ogni forma di odio o di istigazione all'odio e il disegno di legge di cui stiamo parlando contiene questi principi, ma anche altro, come vere e proprie storture, che addirittura vanno a coinvolgere negativamente i minori, i bambini e le famiglie: questo è ciò che ci preoccupa. Vedete - mi rivolgo a quella parte - arrivo da un paese piccolo dell'entroterra ligure, dov'è nato e sepolto Sandro Pertini, il Presidente partigiano,

Probabilmente, se fosse in quest'Aula, con quello che ha fatto e con il contributo che ha dato al nostro Paese, Pertini sarebbe qui a combattere le vostre storture. Non sarebbe qui contro i valori della vita naturale, quella che il Creatore ci ha dato, quei valori su cui, grazie ai sacrifici di molti, è fondata la nostra libera società. Pensateci cercate di riflettere ricordando il passato, perché è arrivato il momento e c'è la possibilità di fare retromarcia in autotutela rispetto a contenuti che non vanno bene e che, in coscienza, anche voi stessi non condividete, sui quali è possibile trovare una via d'uscita e una soluzione: è ciò che noi perseguiamo.

interrotto e dialogato con altre parti. State tranquilli e sicuri che, come sempre, il dibattito viene tutelato nei confronti di tutti. Quindi non c'è bisogno di

Presidente, che basta andare a rivedere le cronache; ho fatto riferimento a fatti veri. La ringrazio anche per il tempo che è stato oggetto di questa interruzione. Credo che tutti insieme

su un binario importante. Sono costretto, anche per il ruolo che ricopro e perché questo purtroppo è l'unico palcoscenico che consente di farlo, a

pagano per svolgere un'attività a cui mediamente è collegato circa lo 0,8 per cento del PIL nazionale. Vi assicuro che non fa piacere sentirsi dire tutti i giorni quello che sto per dire. Leggo, perché è tutto certificato da striscioni, manifesti, video e trasmissioni televisive (in alcuni casi anche mamma RAI si è schierata dalla parte dell'odio): dell'odio): "Siete dei vermi ignobili"; "Fate schifo"; "Sono crepati 41 assassini: grazie per essere morti, soprattutto quelli giovani"; "Vogliamo i vespasiani sulle loro tombe". Sto parlando di manifesti e striscioni che vanno di moda in questo Paese nell'ultimo periodo. Adesso arrivo a spiegarmi meglio, caro Simone: "Cacciatore e pescatore, stessa stesso odore"; "Quando un cacciatore muore, noi brindiamo a tutte le ore" (affisso in una città sotto forma di manifesto funebre);

"Dei cacciatori morti non ce ne frega niente"; "Il cacciatore è un uomo di m. e devono morire tutti"; "Il cacciatore buono è solo quello morto", "Cacciatore? Tre metri sotto terra". Due giorni fa, a Tradate, c'era un fantoccio impiccato con il richiamo a chi pratica quel tipo di attività. Qualche anno fa - chiudo e poi riprendo il filo del discorso discorso - quando morì il Presidente del Consiglio regionale del Trentino, per un infarto durante una battuta di caccia, apparvero manifesti di gioia per la sua morte. Credetemi che non fa piacere vedere giornalmente violenti atti vandalici, non uno qua e uno là, ma costanti e spalmati nel Paese, da parte di animalisti estremisti che entrano nelle proprietà private e distruggono strutture rurali autorizzate. Ebbene, tutti questi italiani, circa 600.000 (con le loro famiglie), subiscono in silenzio queste cose, perché non ne avete mai sentito parlare. *(Applausi)*. È questo il motivo per cui sembra che io stia divagando, rispetto invece all'odio e all'istigazione all'odio. Ma perché nessuno di voi ne parla? Forse perché a una certa parte politica va bene così? Non ho mai sentito nessuno recriminare o fare riferimento ad azioni di odio e di discriminazione o ad atti violenti che costantemente e giornalmente avvengono nel nostro Paese. Forse magari - nessuno si offenda, perché questo è il mio pensiero e credo di poterlo esprimere liberamente qui - perché i mandanti spirituali di quest'odio siedono anche all'interno dell'Aula?

ogni tanto serve qualcuno che ricordi all'opinione pubblica queste cose e che tenga in considerazione che il mondo della ruralità e i diritti di chi paga tasse regionali e governative per svolgere un'attività

esercito, ricordo a me stessa e all'Assemblea che abbiamo costituito una Commissione esattamente per indagare e sottolineare tutte le pratiche di odio. Lo abbiamo ritenuto

Se devo difendere oggi le donne, sotto il profilo della prevenzione di alcuni episodi violenti nei loro confronti, le definisco? No, non ne ho la necessità. ho la necessità. Vorrei ricordare un episodio che mi è capitato trent'anni fa, appena entrata in vigore la legge sulla transizione sessuale.

La consulenza tecnica che era stata disposta sosteneva che non era matura, perché non aveva fatto attività che potessero denunciare la sua effettiva volontà. Riuscii a fare un provvedimento in cui sostenevo che per il sesso - in quel caso, come in questi - non era necessaria un'identificazione,

certamente coinvolgono tutte le definizioni che inserite all'articolo 1. Quali sono? Omofobia e transfobia. Allora perché intestardirsi a voler arrivare a un testo che deve contenere definizioni che non servono ai fini della prevenzione

il nostro sistema penale ritiene che, se istigo la Presidente ad ammazzare un suo amico, ma lei non lo fa, non sono chiamato a rispondere dell'istigazione che ho commesso. Ciò perché l'istigazione a delinquere non è punita, fin dal codice Rocco, ossia quello fascista. E voi volete punire l'istigazione a delinquere.

ed è una cosa chiara e corretta. Quindi immaginate di andare a tradurre questi principi nel testo al nostro esame. Sarebbe perfetto.

perché chi era presente nella passata legislatura, come il senatore Cucca, che era membro della Commissione giustizia, sa che avevamo individuato una formulazione che trovava d'accordo tutti, compreso il Partito Democratico.

comunque punito, ve ne rendete conto? Subisce una sanzione penale. E questa la chiamate possibilità normale di istigazione a un comportamento che non incide sull'opinione?

ho tentato, facendo uno sforzo di interpretazione, di modificare quelle stesse norme in base alla regolarità, alla legge. Questo significa fare ciò che tutti dovremmo,

approntare tutti gli emendamenti, ma, se ci mettiamo a discutere, in due o tre ore riusciremmo a produrre un testo corretto. Non lo volete fare? Significa che volete colpire l'opinione di qualcuno. Questo è tutto.

Allora, cerchiamo di fare la correzione esatta. Questo è l'unico modo per poter ragionare in termini di comportamento coerente con la nostra funzione. Se non lo facciamo, vuol dire che vogliamo abusare,

Dobbiamo avere il coraggio di intervenire per rendere effettiva la sanzione che si vuole introdurre.

al fine di sgombrare il campo da ogni equivoco, voglio dire con forza che, per il sottoscritto, ognuno è libero di amare chi vuole e che, ogni qualvolta si manifestano gesti di intolleranza nei confronti di tutte le minoranze, questi vanno condannati e puniti severamente. E se qualcuno le offende o aggredisce, è solo un cretino e come tale va punito. Fatta questa premessa, dico: togliamo i bambini e le scuole dalla legge.

Per alcuni, ad esempio, i bambini in tenera età devono essere educati su quanti e quali siano gli orientamenti sessuali esistenti, così cercando, a mio avviso, di manipolare la loro crescita emotiva, che, per fortuna, avrà il suo decorso naturale durante la crescita. Sarà allora, una volta cresciuti, che lo Stato dovrà intervenire, mettendo loro a disposizione ogni possibile forma di aiuto psicologico, emotivo ed economico, affinché il disagio svanisca, garantendo a tutti il proprio posto.

prima e ogni forma di intolleranza su sesso, razza, disabilità e religione. *(Applausi)*. Non si può affrontare un problema attraverso una norma penale. Sarebbe come dire che non sappiamo bene come affrontare il problema, per cui lo faccia pure un giudice. Che poi è come dire che ti condanno, tanto poi c'è l'appello; semmai, poi c'è la Cassazione e, se poi sarai assolto, chi se ne frega se nel mentre sei stato alla gogna per dieci anni. Troppa è la discrezionalità nell'interpretazione della norma. Questo modo di risolvere il problema non può mai essere la vera soluzione. È evidente come questo possa incidere sulla libertà di opinione - mi sembra chiaro - lasciando uno spazio ampio, anzi amplissimo, alla discrezionalità dell'organo giudicante. Non lo condivido, signora Presidente, soprattutto oggi, quando il dibattito sulla giustizia è quanto mai acceso. Se l'obiettivo è una giustizia più giusta, lo spazio per la discrezionalità dev'essere sempre più sottile, mai più ampio. Lavoriamo sulle aggravanti, come hanno ben ricordato i miei colleghi della Commissione giustizia e con loro molti altri colleghi in modo trasversale. Bene poi ha fatto il presidente Ostellari a ricordare i tempi con i quali si è affrontata la legge in Commissione giustizia al Senato, sgomberando il campo dalle posizioni strumentali di chi voleva evitare il confronto a favore dell'arrocco ad ogni costo. Al presidente Grasso, che non è in Aula oggi, ma, replicando al presidente Ostellari, ha esordito parlando di verità, come se ne fosse l'unico custode, dico che lui racconta la sua verità e che l'astio con il quale si è rivolto al presidente Ostellari fa trasparire in modo evidente quanto ancora sia turbato dalla sua mancata elezione a quel ruolo: oggi sarebbe il il caso che la metabolizzasse, cercando alla sua sinistra le ragioni di quella sconfitta. *(Applausi)*. Il fronte di coloro che vorrebbero modificare la legge, per renderla di tutti, non solo di alcuni, e fare in modo che questo non sia un manifesto ideologico, si fa sempre più ampio, anche tra le fila del centrosinistra. I distinguo sono ormai davvero molti. A questo proposito, voglio citarne uno solo, riprendendo una frase, o poco più, estrapolata da un'intervista molto più ampia, che mi ha convinto e commosso allo stesso tempo. La frase è del senatore Faraone, che, intervistato sul disegno di «Proprio perché deve colpire gli abusi, i crimini, le prevaricazioni, deve essere scritta bene e non dare adito a dubbi interpretativi. Questo il compito che dobbiamo affidare alla legge. Punto. Vogliamo allargare i diritti o accontentarci della bandierina? Io non ho dubbi su cosa fare». Invito tutti a leggere la sua intervista, rilasciata come senatore, ma come padre innanzitutto. Anche per le ragioni molto ben esposte dal collega abbiamo più volte ripetuto al Partito Democratico che servirebbe un confronto serio sul tema, togliendo i temi divisivi e lasciando l'impianto di una legge che tutti siamo pronti a votare. Purtroppo ogni singola apertura e ogni singola proposta fatta da noi, ma anche da molti altri, affinché si approvi la legge con il voto di tutti, si sono inesorabilmente scontrate con il muro eretto dal segretario Letta, che ci fa pensare ci sia una scelta più strategica che di buon senso. Il suo posizionamento mi induce a fare un paio di riflessioni. La prima è che, alla fine di questi mesi di scontri sul testo, forse sia arrivato a metabolizzare, a comprendere e a realizzare che, così com'è, esso non sia il migliore possibile, per cui il suo arrocco consapevole determinerà la morte del disegno di legge in oggetto, ma nel contempo darà soddisfazione a quell'area di sinistra del suo partito e della sua alleanza, evitando una guerra interna e spostandola al di fuori del perimetro del centrosinistra. Contento lui, buona fortuna. La seconda: nessun accordo per compiacere Conte, l'uomo dei mille carpiati, che, secondo l'Enrico da Parigi, è l'alleato giusto per sconfiggere questo centrodestra a trazione leghista, tralasciando, a mio avviso, due piccolissimi particolari. Il primo è che la fascia di mercato a cui si rivolgono è esattamente la stessa (quindi, buona fortuna) e il secondo è l'errore di sottovalutare l'ambizione dell'ex avvocato del popolo. Ma si sa: ai posteri l'ardua sentenza.

"Papà sei un X", mi hanno detto i miei figli. Noi senatori siamo definiti dalle nuove generazioni e dagli *influencer* di turno come *boomer* o generazione X,

che si chiamano generazione Z, che sono i veri nativi digitali, quelli che si confrontano sul *web*. Noi *boomer* o generazione X, secondo i giovani, siamo coloro che etichettano, che definiscono le persone in categorie; loro invece le identificano come persone, non più tra maschi e femmine perché una persona può sentirsi anche un'altra cosa. Poi, magari, i nuovi giovani possono arrivare a pensare che la nostra posizione sul disegno di legge Zan sia giustificata da poter essere liberi di insultare le minoranze, senza essere puniti per questo e chissà quale altra nefandezza. Guardate, giovani e rivoluzionari - lo dico ai ragazzi, e lo dico anche ai miei figli, in realtà - lo siamo stati tutti, chi più chi meno. Ma sono certo che la vera stella polare che dovrebbe guidare le persona di tutte le età sia quella del rispetto per ogni differenza, sia essa di genere, di razza, eccetera eccetera. Definire Definire un maschio o una femmina, un omosessuale, una lesbica, un cattolico, un ebreo, un musulmano non è una discriminazione per nessuno, ma solamente una banale definizione, utile a sottolineare quelle differenze che ci sono e che tanto si vogliono difendere; ma con questa legge, così com'è, ciò non potrà mai accadere. Alla generazione Z dico che sono cresciuto rispettoso degli altri, con le mie idee consolidate nel tempo: come tutti, da ragazzo pensavo di avere ogni verità in tasca, mi sentivo forte e spavaldo, ma mai e poi mai ho sentito la necessità di insultare, di ghettizzare le persone per i loro orientamenti sessuali, religiosi o altro. La vera differenza tra i *boomer* e la generazione Z sta nell'esposizione diversa delle informazioni.

Su temi come questo - proprio perché di sicuro siete meno ignoranti di noi o lo siete meno di quanto lo eravamo noi - usate questa mole di informazioni per confrontarle tra loro, matchatele; ascoltate tutte le tesi in campo non lasciatevi intimidire dall'opinione di coloro seguiti sui *social*. Anzi, mettetele in discussione perché spesso - non sempre evidentemente - dietro si celano meno nobili intenzioni. Ricordatevi che è solo una questione di tempo e prima o poi *boomer* lo diventerete anche voi. Mi piace citare una frase di chiusura di un noto programma radiofonico in onda nel pomeriggio: tutti hanno il diritto di avere un'opinione, ma tutti hanno il dovere di averla informata. Per questo dico che poco mi importa di quale sarà l'opinione, purché sia figlia di questa premessa. Concludo con un auspicio, signora Presidente, del tutto personale, credetemi. Come è accaduto per questa legge, il confronto con i miei figli è stato acceso - devo ammetterlo, molto acceso - ma possa esserci sempre e a prescindere dall'argomento e dalle rispettive posizioni, a volte importanti e complicate come in questo caso, ma sempre con un unico obiettivo: offrire loro la possibilità di avere la possibilità di avere la propria opinione senza imporla né come genitore né tanto meno come legislatore. *(Applausi)*. PRESIDENTE.

viviamo un momento storico in cui i sacrifici fatti dai giovani sono completamente differenti da quelli della nostra epoca o dell'epoca dei nostri genitori. Si combatte meno e si ottiene tutto con troppa facilità. Questa mancanza di dedizione porta le nuove generazioni ad abbandonare tutto alle prime difficoltà. In Italia la quota di popolazione con titolo di studio terziario continua a essere molto bassa rispetto all'Unione europea, ma per fortuna non sempre è così. In concomitanza con la vittoria dei calciatori azzurri ai campionati europei è emersa una giovane atleta. È di lei che voglio parlare: ha dimostrato *mens sana in corpore sano* e che prendersi cura del proprio corpo, condurre una vita sana per avere una mente lucida, attenta a sfruttare al 100 per cento le doti cognitive, può portare a risultati eccezionali. Questo è successo a lei. Si chiama Dalia Kaddari. Nasce a Cagliari il 23 marzo 2001 da madre sarda e padre marocchino che da trent'anni vive in Sardegna e fa il commerciante. L'integrazione in Italia è possibile. Rispetto delle regole, assimilazione delle leggi italiane, diritto all'istruzione e al lavoro, esempio di perfetta integrazione: Dalia si fa notare; è bellissima, è stata miss Quartu, città dove risiede, ed è velocissima, campionessa italiana dei 200 metri. Inizia in tenera età con il basket e poi i suoi istruttori capiscono il suo talento per l'atletica. La *sprinter* italiana sarda delle Fiamme oro, gruppo sportivo della Polizia di Stato, conquista ancora *juniores* la prima maglia tricolore, che consolida la sua seconda posizione nella lista italiana della categoria. È stata seconda sugli 80 agli studenteschi del 2015 e così di seguito. La sua è stata una collezione di trofei: l'ultimo, in ordine cronologico, è la medaglia d'argento conquistata in Polonia agli Europei a squadre. L'atleta delle Fiamme oro ha fatto registrare il primato personale sui 200 metri al Golden Gala, che vale anche il *record* europeo *under* 23, il terzo crono di sempre per un'italiana sui 200 metri piani femminili, e ha conquistato la medaglia d'oro. Quando il *premier* Draghi ha posato per la foto ufficiale con la Coppa europea vinta dagli Azzurri, ha voluto Dalia al suo fianco. Dalia, una ragazza acqua e sapone, sempre sorridente, un esempio di costanza e determinazione, alle sfilate ha preferito lo sport, la competizione, il sacrificio; la campionessa dei 200 metri, vero orgoglio di Sardegna, la terza italiana più veloce di sempre. Che sia Dalia, Presidente, un esempio: ha appreso il sacrificio, il rispetto per la famiglia e per il prossimo, l'amore per lo sport, conduce una vita sana per sfruttare al meglio la capacità e dare il massimo a scuola e all'università.

Carlo Giuliani è stato ucciso a Genova in piazza Alimonda, in uno dei giorni più bui per la nostra Repubblica. Quella piazza dove morì venne ribattezzata dai suoi compagni "Piazza Carlo Giuliani, ragazzo", perché Carlo era un ragazzo di ventitré anni e condivideva i sogni, le speranze, la rabbia di tanti della sua e della nostra generazione; un ragazzo di ventitré anni colpito da un altro ragazzo di venti anni, vittime entrambi; due ragazzi che si fronteggiavano quando in una democrazia non sarebbe mai dovuto succedere. Non dovrebbero esistere, in una democrazia, barricate e mai avrebbero dovuto fronteggiarsi come nemici manifestanti e Forze dell'ordine; due ragazzi per entrambi i quali proviamo dolore, nonostante il destino diverso e le diverse responsabilità. In quei giorni, vent'anni fa, a Genova c'era il G8, il *meeting* dei grandi del pianeta, a Genova si diedero appuntamento migliaia di ragazze e di ragazzi da ogni continente per chiedere un mondo più giusto. Quei ragazzi non avevano niente a che spartire con le tute nere dei *black bloc* che saccheggiarono e devastarono la città senza che nessuno li fermasse. Quei ragazzi volevano far sentire la propria voce ai potenti del mondo, ma vennero zittiti da una repressione cieca. Fu un abuso di potere, un esercizio di violenza contro un'intera generazione. Molti che erano lì non si ripresero mai da quello che subirono, da quello che avvenne in quelle vie, in quelle piazze, nell'orrore della notte della scuola Diaz e della caserma Bolzaneto. Quei ragazzi vennero torturati da chi avrebbe dovuto tutelarli, come accertato dalla magistratura. Fu tortura, come disse anni dopo il capo della Polizia Franco Gabrielli. Fu la notte in cui il nostro Stato di diritto venne stracciato da chi avrebbe dovuto difenderlo, da chi aveva giurato sulla nostra Costituzione. Penso che dobbiamo ricordarlo, penso che la politica debba farlo, in particolare chi, come noi, crede nella funzione civile e democratica delle nostre forze di sicurezza. Mai più servitori dello Stato infedeli, mai più violenze e arbitri, mai più fatti come quelli di Genova o - è cronaca di questi giorni - fatti come quelli di Santa Maria Capua Vetere

Signor Presidente, tutta Europa in questi giorni è stata attraversata da un'insidiosa perturbazione atmosferica, l'ennesima; in Germania una vera catastrofe: 165 vittime e disastri tutto attorno. Ormai la frequenza di questi fenomeni atmosferici ha raggiunto livelli da guerra permanente. L'allarme fu lanciato già nel Summit della Terra di Rio de Janeiro, nel giugno del 1992, in cui si capì che le conseguenze di un sistema produttivo e di stili di vita inconciliabili con l'equilibrio naturale avrebbero causato fenomeni disastrosi come quelli di questi giorni. Il mio intervento oggi vuole essere la voce dei tanti imprenditori e abitanti dei territori colpiti dalle svariate calamità naturali che tutti noi, in momenti diversi, abbiamo ascoltato e vissuto. Vivo è il grido di aiuto che ieri si è levato dalla provincia di Foggia, da Rignano Garganico, da San Marco in Lamis, da San Giovanni Rotondo, il mio territorio, che ha vissuto ore di grande paura e ha rischiato anche di contare vite umane; pericolo per fortuna scampato, grazie ai coraggiosi soccorsi. Ora si è alla conta dei danni. Tante sono le aziende agricole pesantemente danneggiate e i raccolti distrutti; danni ingenti anche al manto stradale. Urgenti sono gli interventi di ripristino ora necessari. Ieri tutti erano in campo, nel tentativo di salvare il salvabile: Protezione civile, Vigili del fuoco e comuni cittadini; tutti sono intervenuti al fianco dei sindaci, sempre in linea nell'affrontare ogni emergenza; tante ore, senza sosta; uomini spinti da spirito di servizio e passione, che tutte le volte ne fanno degli eroi. A loro va il mio ringraziamento incondizionato. Ieri sono accorsa anch'io, appena appreso della gravità della situazione. Per me è stato importante condividere quei momenti, importanti la solidarietà e la condivisione del carico dei problemi per trovare insieme le soluzioni possibili. Nel cuore e nella mente ho quelle immagini, quei volti che ora condivido con voi, perché tutti dobbiamo far sì che la ripresa sia rapida e reale. Indispensabile è il lavoro di una politica concreta e responsabile, a tutti i livelli, ma anche di operatori dei vari settori onesti e rigorosi. Mi auguro che tutto questo si concretizzi presto.

le intense piogge che il 14 e il 15 luglio hanno interessato Germania, Olanda, Belgio e Lussemburgo hanno causato catastrofiche alluvioni con gravi perdite di vite umane e danni per svariati miliardi di euro. Un territorio di 50.000 chilometri quadrati è stato sconvolto: Schuld, Insul e Sinzig distrutte peggio che in un bombardamento. Ci stringiamo in un abbraccio solidale e fraterno con i popoli colpiti, non solo virtuale, dato anche l'invio della nostra Protezione civile. In tanti hanno associato l'accaduto a fenomeni meteo estremi, innescati dal surriscaldamento globale dovuto ai gas serra di origine antropica. Nella realtà, allarmi ignorati, urbanizzazioni intorno ai fiumi o finanche dentro, imbrigliandoli, deviandoli, tombandoli, oltre a pesanti lavorazioni agricole sono il *mix* che, unito al cambiamento climatico, ha trasformato un'intensa pioggia in catastrofe. Le inondazioni erano previste, ma sembra che gli allarmi del servizio di monitoraggio siano stati ignorati o sottovalutati dalle autorità locali. Afferma Violo, presidente del Consiglio nazionale dei geologi, che il problema non è la particolare intensità delle precipitazioni, quanto la risposta idrologica e morfologica dei territori, urbanizzati senza adeguata pianificazione. ricerche, che dice che, agli eccessi di cementificazione e di estrazione, la natura risponde disintegrando argini inadeguati e riprendendosi i suoi spazi. Quando si progetta un'opera, bisogna oramai tenere in conto i futuri scenari di deriva climatica. Conosciamo le cause: aumento dei gas serra; deforestazione; agricoltura e allevamento non sostenibile. Possiamo, quindi, fare qualcosa per ridurre gli effetti dannosi di questa attività. Urge poi prevenire, mitigare e ridurre il dissesto idrogeologico e adattare i territori e le costruzioni al nuovo clima. Occorre ripristinare gli ecosistemi fluviali e recuperare gli spazi che con devastanti conseguenze abbiamo rubato ai fiumi, in linea con la strategia europea per la biodiversità, che impegna gli Stati a rinaturalizzare e riconnettere almeno 25.000 chilometri di fiumi entro il 2030. Urge una vera e propria ecologia integrale.